Signor Presidente, è con rammarico che devo comunicare a lei e all'Assemblea che, a causa del brevissimo tempo a disposizione per l'esame di questo disegno di legge, non è stato possibile completare - devo dire nemmeno iniziare - la discussione nelle Commissioni riunite e pertanto oggi ci presentiamo in Aula senza il mandato al relatore. Colgo l'occasione - non è la prima volta - per manifestare il mio disagio come Presidente della 1a Commissione nel dover registrare che, purtroppo, questi

e quindi comprendiamo le ragioni che, a volte, possono portare a una compressione così drastica dei tempi di esame e di discussione. Tuttavia, signor Presidente, di far presente al Governo che questa non può diventare la regola, perché è una compressione inaccettabile delle prerogative del Parlamento. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Balboni, il disegno di legge n. 829, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento Dichiaro aperta la discussione generale. Signor Presidente, colleghi e colleghe, le parole del presidente Balboni non avrebbero necessità di essere commentate, perché sono parole che esprimono una consapevolezza grande di quanto da tempo il Partito Democratico va lamentando. Non posso quindi non associarmi

anche alla maggioranza e - ne sono convinta - farebbe molto bene anche a chi governa. Ascoltare e provare a confrontarsi sui provvedimenti è una scelta, un'opzione di saggezza. Siamo abituati e ci stiamo abituando, ma continueremo a denunciare le presunte urgenze a cui il Parlamento viene costretto di volta in volta, votare la fiducia e a dare vita a quello che non si può non definire un monocameralismo di fatto, perché i provvedimenti vengono discussi,

vada portato all'attenzione dei Presidenti delle due Camere e anche della Presidenza della Repubblica. È un modo di legiferare e di governare che non può essere accettato. Mi lasci aggiungere, Presidente, che avendo vissuto da Sottosegretaria la pandemia, non posso dimenticare le denunce scandalizzate che accompagnavano le urgenze, che credo non si possano non definire tali. Quando parliamo infatti di una pandemia, come è stata quella del Covid-19, non si può non dire che quella era davvero un'emergenza, che ci costringeva anche a tempi accorciati nelle decisioni e nell'assunzione di norme, che servivano immediatamente.

che non si è voluto cambiare in nulla e non si vuole affrontare un problema, che è quello di non dare più il tempo, a noi parlamentari, di esercitare i nostri fondamentali nostre prerogative, che prima di tutto prevedono una discussione e un confronto nelle sedi opportune, a cominciare dalle Commissioni. Capita di continuo e ormai ci stiamo, nostro malgrado, abituando - ma, come ho detto, continueremo a denunciarlo con sempre maggiore vigore e veemenza - a una mancanza di confronto con la maggioranza e a doverci esprimere solo con dei sì o dei no,

si va dall'università, alla salute, alla vigilanza, alle materie prime, alla cultura, alle malattie infettive e all'abbattimento degli animali, alla medicina preventiva, alle olimpiadi di Cortina d'Ampezzo,

In questo modo viene completamente disattesa l'applicazione dell'articolo 97 della Costituzione, che vuole siano assicurati il «buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione», che devono essere l'obiettivo primario, soprattutto del Governo. Anche qui duole misurare la distanza enorme tra le parole pronunciate e la propaganda che è stata consumata sul valore della pubblica amministrazione, su quanto conti una pubblica amministrazione valorizzata, efficiente e funzionante, e quanto invece oggi manifestiate un'assoluta distanza e persino una mancanza di rispetto nei confronti di quello che dovrebbe essere il motore dello Stato. Mi pare che infarcendo questo disegno di legge di varie ed eventuali, non si arrivi a toccare alla fine nessun punto saliente e che si vogliano solo agitare un po' le acque, promettendo cambiamenti che di fatto non ci sono e non ci saranno. Leggendo il contenuto del provvedimento si ha l'idea, lo ribadisco, di una gran confusione, di un lavoro portato avanti in maniera poco organica e di avere voluto solo superficialmente occuparsi di un settore strategico per il futuro del Paese. Almeno per noi parlamentari del Partito Democratico la pubblica amministrazione è ciò che rappresenta un tema nevralgico per il nostro Paese. Come si può pensare di non affrontare seriamente un tema come questo? Ci sono più di tre milioni di lavoratrici e lavoratori a cui è affidata quotidianamente l'erogazione di servizi per la qualità della vita di cittadini e imprese e non parliamo di questioni astratte, ma di attività che riguardano davvero la vita di ogni cittadino italiano. Se volessimo fare un riferimento semplice da capire, viste le ultime incresciose vicende che hanno riguardato da vicino l'Italia, colpita dalle alluvioni e piegata dagli incendi, possiamo riferirci agli uomini e alle donne impiegati nei Vigili del fuoco. Ma io ho in mente le tante migliaia di di dipendenti pubblici che ogni giorno compiono il proprio dovere e avrebbero bisogno di trovarsi in un contesto efficiente, che valorizzi il loro lavoro. C'è anche un grande bisogno di cambiamento di competenze. Queste ultime settimane di incendi e alluvioni hanno messo a dura prova il Paese e sono stati impegnati senza sosta Vigili del fuoco e Forze dell'ordine, per tutto il giorno, e così i Comuni e i loro dipendenti, lavoratori che, appunto, svolgono con abnegazione impagabile il proprio dovere. A loro - permettetemi di farlo in questa sede - va il nostro ringraziamento e, ribadisco, il rammarico per non vederli davvero messi al centro di un'azione di valorizzazione. Anche alla luce di tutto questo, è innegabile che dalla pubblica amministrazione non passi, appunto, solo l'erogazione dei servizi, ma la realizzazione di quello straordinario piano di investimenti che si chiama Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con chi pensate di realizzare il PNRR se non con i dipendenti pubblici? Il PNRR, lo sappiamo, è un pacchetto di 750 miliardi di euro concordato con l'Unione europea in risposta a una crisi gravissima che ha colpito il nostro Paese e per tornare alla pubblica amministrazione ci si è in pratica dimenticati, in questo provvedimento, che siamo qui a discutere che cosa sia e di che cosa abbia bisogno. Voglio ricordare che è proprio dalla pubblica amministrazione che oggi passa anche un pezzo di sviluppo del nostro Paese, un pezzo molto importante. Senza una pubblica amministrazione davvero efficiente e messa nelle condizioni di lavorare, anche grazie a cambiamenti e riforme necessarie, noi non vedremo ripartire lo sviluppo dell'Italia. Abbiamo bisogno di misure concrete per trasformare il settore pubblico in un vero e proprio motore dello sviluppo.

con un ultimo cenno alle parole improprie che il ministro Crosetto ha pronunciato l'altro giorno su un Parlamento che non lavorerebbe abbastanza. Ecco, a me pare che quello che sta succedendo qui oggi sia la replica e la risposta migliore che gli italiani devono conoscere su quale sia il problema di questo Parlamento nella sua capacità di lavorare e di lavorare con efficacia; quella che i cittadini che ci hanno eletti e mandati qui a rappresentarli chiedono ed esigono.

Ovviamente il fatto che il Senato non ne potesse discutere il merito dice non solo dell'eccessiva decretazione d'urgenza che si utilizza, ma anche delle modalità con cui si sta affrontando il rapporto tra il ruolo del Governo e il potere legislativo del Parlamento, che sempre più viene messo in discussione. In qualche caso potremmo dire che ci sentiamo umiliati nella nostra funzione di senatori e di senatrici nell'affrontare in questo modo il processo decisionale e legislativo. Vale poco

molta attenzione a moltiplicare i ruoli di direzione e le direzioni dei Ministeri, la totale disattenzione allo stato davvero difficile in cui versa la nostra pubblica amministrazione. Io non so se abbiamo avuto la pazienza di guardare qualche numero rispetto a quello che sta succedendo nella pubblica amministrazione, ma vorrei per esempio dire al ministro Fitto, che ci diceva che bisogna tagliare delle parti del PNRR perché non sappiamo se siamo in grado di rendicontarle, che se non si mette mano alla struttura e alla quantità di lavoratori e di lavoratrici nella pubblica amministrazione continueremo a non saper rendicontare, perché non potremo farlo. *(Applausi)*. Da questo punto di vista il tema non riguarda solo il PNRR, perché qualunque bando, qualunque finanziamento europeo, qualunque accesso a quelle risorse richiede di avere le figure tecniche nelle amministrazioni che siano in grado di farlo. farlo. Non vanno quindi bene due decreti-legge (ma non sarebbe andato bene neanche uno solo) se sono solo finalizzati a mettere qualche toppa senza affrontare invece le questioni fondamentali della nostra pubblica amministrazione,

ruolo e nella loro capacità di dare risposte. Credo che sia sotto gli occhi di tutti ciò che sta succedendo nella sanità, dove non solo l'anzianità media del personale è troppo alta e non permette di governare le sfide che ci presenta la situazione attuale, ma c'è anche e soprattutto una demotivazione che riguarda le modalità del lavoro, la quantità delle persone che possono lavorare e le risposte che si devono dare. La Presidente del Consiglio ci dice che lei sarebbe contro il salario minimo, che pure in tanta parte della pubblica amministrazione sarebbe fondamentale, se pensiamo ai processi di esternalizzazione e di appalto che caratterizzano questo settore *(Applausi);* tuttavia, anche se non guardiamo a questo elemento, ci dice che non si può fare, perché bisogna valorizzare la contrattazione. chiederle perché questi due decreti-legge, uno dopo l'altro, non hanno mai visto la partecipazione delle parti sociali e la discussione con loro; forse perché quelle parti sociali avrebbero detto che il problema non era nel numero delle direzioni in questo o quel Mistero, ma negli organici, nei contratti, nelle qualità professionali. Approfitto però di questo elemento che riguarda appunto il rapporto con le parti sociali e la contrattazione per dire che questo secondo decreto-legge sulla pubblica amministrazione è anche caratterizzato dalla furbizia dell'ultimo minuto. Mentre era in corso alla Camera l'ultima notte di discussione sugli emendamenti, il Governo e il partito di maggioranza relativa hanno deciso di accogliere una "scialuppa", che casualmente veniva da Italia Viva, per decidere di cambiare l'esito di circa 30 milioni di finanziamenti nei prossimi anni, che passano dal comitato denominato "Previdenza Italia", ad Assoprevidenza. So che probabilmente appassiona pochi discutere di previdenza complementare, ma forse sarebbe bene che anche qui qualche numero provassimo a ricordarcelo. Il nostro Paese ha passato alla fiscalità generale circa 21 miliardi di contributi che le aziende dovrebbero pagare per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti. Negli ultimi mesi - Governo Draghi prima, Governo Meloni poi - circa altri 13 miliardi sono passati alla fiscalità generale per intervento sul cuneo fiscale. Quelli, almeno, sono a vantaggio dei lavoratori e sono stati un primo sollievo rispetto ai problemi dell'inflazione e della scarsità dei salari. Tutto si può dire, quindi, tranne che le politiche non governino ampiamente il tema della previdenza, forse non nella direzione che sarebbe coerente a un sistema contributivo quale quello che abbiamo. Ma è esattamente perché abbiamo un sistema contributivo che la previdenza complementare è diventato un elemento essenziale per la condizione dei lavoratori. la previdenza complementare può essere fatta in due modi: con gli accordi contrattuali, che hanno un vantaggio diretto per i lavoratori non solo perché avviene sulla loro retribuzione e sul loro trattamento di fine rapporto, ma perché c'è una quota che le aziende mettono ad aumentare la capitalizzazione, oppure con il sistema privato assicurativo, con i fondi chiusi, con i PIP, in tutte le varie forme con cui le assicurazioni generano profitto sul nostro futuro destino previdenziale. Ebbene, avremmo bisogno di ampliare la previdenza contrattuale, avremmo bisogno di dare più risposte ai lavoratori e alle lavoratrici, di darle a quei lavoratori e a quelle lavoratrici, agli artigiani, alle piccole imprese, dove c'è un bisogno di informazione. Per questo era nato, insieme alle parti sociali, il comitato "Previdenza Italia". Perché si sia deciso, invece, di finanziare le assicurazioni di un'associazione privata resta un mistero, ma forse è uno di quei misteri di cui poi chi pagherà il prezzo saranno i lavoratori e le lavoratrici.

i Governi precedenti. Ricordiamo le critiche al Governo Draghi, quando si diceva che si continuava a decretare d'urgenza e a mettere la fiducia. Ebbene, voi avete già superato abbondantemente questo *record* solo in pochi mesi.

lo svuotamento delle prerogative essenziali del Parlamento, che sono quelle del confronto, dell'ascolto, del dibattito, che farebbero bene sia al Governo che al Parlamento tutto.

Anche ieri i giornali hanno dedicato tantissime pagine a questo tema, evidenziando un buco di 15 miliardi di euro nella sanità. Significa mandare all'aria un sistema sanitario pubblico, nazionale e universale, che è un fiore all'occhiello in tutto il mondo. Allora perché non trovare risorse dove realmente c'è bisogno? Questa sicuramente non solo è una priorità, ma noi avevamo anche indicato - come facciamo di solito, essendo un'opposizione costruttiva e propositiva - dove reperire quelle risorse, ma non siamo stati ascoltati. Questo avviene un po' in tutti i settori che avete cercato di mettere assieme in maniera confusa in questo provvedimento, per esempio sulle assunzioni. Quale meritocrazia? Non ne abbiamo discusso abbastanza, perché non c'è stato il tempo, ma anche questo atteggiamento non ci è piaciuto assolutamente. Nessuna meritocrazia anche sul tema delle assunzioni. Sullo sport, all'articolo 34, che dovrebbe regolamentare l'ambito dei processi sportivi, si prevede che il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguino i propri statuti con l'obiettivo di rendere applicabili le penalità solo una volta che la sentenza sia passata in giudicato. Questo riguarda, nei provvedimenti davanti alla giustizia sportiva, l'impugnazione di sanzioni o di penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare, per esempio, la classifica finale delle competizioni a squadra. a squadra. Da sportiva, lasciatemi dire che la bontà della finalità della norma è svilita da un atteggiamento che, a mio avviso, va a violare l'autonomia del CONI e dell'ordinamento sportivo nella sua interezza. Questo Governo - lo sappiamo - porterà sicuramente a ricorsi all'autorità giudiziaria e alla Corte costituzionale, che peraltro si è già espressa in maniera netta anche in merito a questo. a questo. Negli articoli 38 e 39, che riguardano i giochi di Milano-Cortina 2026, si prevede l'estensione della possibilità di sottoscrivere contratti di lavoro subordinato, senza specificare dei limiti temporali, purché riguardino l'ambito dello svolgimento dei giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2026. Anche qui sarebbe stato opportuno ampliare il numero dei Comuni, perché non si capisce perché alcuni saranno beneficiari e altri no, penalizzando per esempio moltissimo i Comuni lombardi. Potrei continuare così, ma voglio chiudere sul tema della cultura, che a noi sta molto a cuore: intanto sull'App 18 del Governo Renzi, dove non si sono trovate le risorse, quante volte l'abbiamo detto al ministro Sangiuliano? Poi, nelle disposizioni di cui all'articolo 12-*bis*, relative alla fondazione Centro sperimentale per la cinematografia, apprendiamo che si svilisce quella che dovrebbe essere l'autonomia e l'indipendenza della cultura e del cinema. Oltre a sopprimere la figura del direttore generale, viene prevista la nomina del comitato scientifico da parte del Ministro della cultura, composto da sei componenti, il quale si sostituisce anche al consiglio di amministrazione nell'indicazione del presidente. Anche questa noi la consideriamo una vera e propria lottizzazione, così com'è accaduto con la RAI. In conclusione, noi siamo rimasti sempre con un atteggiamento propositivo e abbiamo cercato, soprattutto alla Camera, dove c'è stata la possibilità di un minimo di confronto, di fare proposte emendative che andassero nella direzione di individuare le priorità. Non c'è stato alcun ascolto in questo senso e qui in Senato siamo arrivati a ridosso ormai delle vacanze estive. Quindi mi dispiace, Governo, ancora una volta si è persa una grande occasione per ribadire quanto la sanità, la cultura, il lavoro,

all'interno di questo decreto-legge, che sia stato partorito dalla maggioranza, ma mi risulta piuttosto difficile, un po' per i contenuti e un po' per l'enormità di tempo che ci avete concesso per esaminarlo, cosiddetto PA, passato da queste Aule come un fulmine: ormai ci stiamo abituando. Chiederei almeno la grazia al Governo: se, quantomeno per argomenti, riuscisse ogni tanto a far lavorare tutte e due le Camere, non sarebbe un dispiacere *(Applausi)*; e magari così riusciremmo ad essere un po' meno pungenti nei vostri confronti, poche cose degne di nota e, tra queste, ve ne sono alcune ottenute con ordini del giorno dei miei colleghi, che fortunatamente sono riusciti a lavorare nell'altra Camera:

che è stata salutata con piacere dai sindacati della Polizia, e infatti subito il Governo ha cercato di prendersene i meriti. Complimenti, siete bravi a prendervi i meriti per il lavoro degli altri; davvero, complimenti.

attive del lavoro (ANPAL). Avete cancellato il reddito di cittadinanza, se ne sono accorti tutti; l'avete fatto a dicembre e avevate detto che entro sette mesi avreste messo insieme le politiche attive del lavoro, che gli occupabili sarebbero stati avviati a un corso e che nessuno sarebbe stato lasciato indietro. Ce ne siamo accorti benissimo, infatti all'improvviso è arrivato uno SMS, nessuno ha iniziato alcun corso, le politiche attive del lavoro giacciono dimenticate dalle Regioni, che dovrebbero farle, ma non le hanno mai fatte, neanche quando glielo abbiamo chiesto e gli abbiamo dato i soldi per potenziarsi. Però qualcosa fate: prendete ANPAL e la trasformate. Facciamo il gioco delle tre carte: le funzioni le spostiamo al Ministero, cambiamo nome all'Agenzia, le facciamo fare qualcos'altro, buttiamo un po' di fumo negli occhi e magari nessuno si accorge che non stiamo facendo niente anche se avevate detto di essere pronti. Non ho capito ancora pronti a cosa, però va bene. Che altro? Un altro merito, in realtà, non è del provvedimento, bensì di qualcuno che ci ha aggiunto qualcosa. Stavolta avremmo preferito che non fosse successo, ma, come al solito, i colleghi di Italia Viva riescono a fare le stampelle della maggioranza e, invece di fare l'opposizione, fanno l'opposizione all'opposizione: presentano un emendamento che con il vostro contributo soffia 29 milioni di euro al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare e li regala ad Assoprevidenza, facendo fare a una società a una società *profit* quello che doveva fare l'ente terzo *super partes*. Bravi! *(Applausi)*. Questo nonostante i moniti del Quirinale. Complimenti davvero ai colleghi di Italia Viva e alla maggioranza che gli è andata dietro. Questo emendamento era stato già inserito nel decreto-legge bollette, ma è stato espunto, perché evidentemente a qualcuno non era gradito (giustamente), ma voi ce lo avete infilato di nuovo dalla porta di servizio. Complimenti, davvero. E che dire delle norme sulla Polizia penitenziaria? Nei giorni scorsi, a Torino c'è stato l'ennesimo suicidio di un detenuto, anche tra i lavoratori della Polizia penitenziaria c'è un tasso di suicidi nettamente superiore rispetto a quello della popolazione generale. Lamentano carenze perché l'organico della Polizia penitenziaria, per cui sarebbero previste 45.000 unità, è stato ridotto a 41.000. In servizio in realtà ce ne sono 36.000 che si devono occupare

Lo troviamo infarcito infatti di provvedimenti fondamentali e urgenti per il Paese, come l'aumento del trattamento economico degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri. *(Applausi)*. Sicuramente una cosa di cui c'erano assolutamente

erano tanti gli articoli da valutare in così poco tempo, pertanto mi scuserete. Davvero non avete lasciato indietro nessuno all'interno dei Ministeri. Complimenti! *(Applausi)*. ricordo alcuni decenni fa un partito di maggioranza che urlava contro «Roma ladrona», contro il «magna magna», contro il centralismo. Siamo anche a discutere fuori da quest'Aula di regionalismo asimmetrico e di autonomia e invece potenziate gli apparati centrali. La coerenza è veramente il vostro faro. Bravi! Bravi! Continuiamo così, che andiamo bene. *(Applausi)*. Mi ero dimenticata l'ultima chicca: la peste suina africana. Chi come me arriva dal Piemonte, dov'è scoppiato l'ultimo focolaio, sa bene che è stato un grande problema. Come decidete di contribuire a risolverlo? Con le doppiette per ammazzare i cinghiali. Certo! *(Applausi)*. E anche con una norma per fare in modo poi che la carne di cinghiale ce la mangiamo: mica la vorremo far andare sprecata, giustamente. Riduciamo gli sprechi, è logico. Roma era tutto un «magna magna», ma evidentemente «magnà» è piaciuto pure a voi, soprattutto se si tratta di carne di cinghiale. Bravi!

Presidente, Sottosegretario, Ministro, senza mancarle di rispetto vorrei intervenire dicendo «ancora tu», ma non è il «tu» per utilizzare un linguaggio confidenziale, è che noi

i posti apicali. PA sta per posti apicali, perché voi nei due decreti-legge chiamati PA vi siete solo occupati di garantire, cambiandoli o ampliandoli, per i Ministeri e posizioni che voi avete voluto occupare con forza. Dimentichiamoci che stiamo trattando un decreto-legge sulla pubblica amministrazione, perché questo è tutt'altro. Capiamo benissimo anche la vergogna o l'imbarazzo del ministro Zangrillo, che a breve distanza è costretto a fare due decreti-legge per correggersi o per inserire punti che non erano stati trattati in maniera approfondita o completa. Con il primo decreto, che tra l'altro, come ricordava prima la collega Pirro, qui non abbiamo visto, come non abbiamo visto questo - forse, lo dico ai colleghi, noi non possiamo affrontare i temi della pubblica amministrazione, cioè avete deciso che questo ramo del Parlamento non debba trattare l'argomento l'argomento - avete utilizzato il provvedimento come strumento per occupare i posti dirigenziali e apicali negli enti pubblici e nelle partecipate.

perché non vi accontentate di quello che è già nelle vostre mani e nelle vostre facoltà: siete intervenuti anche a gamba tesa su tutto ciò che invece aveva un principio forte di autonomia, di indipendenza e di creatività. Mi riferisco al gravissimo attacco che avete fatto al Centro sperimentale di cinematografia (CSC), che ci ha molto colpito e rimaniamo stupiti del fatto che non siate colpiti voi. C'è stata una grande mobilitazione da parte delle studentesse e degli studenti, che hanno contestato il metodo e il merito attraverso i quali sono state introdotte modifiche sulla *governance* piacciono da matti: ci mettete sei, sette o otto mesi per rifarle, le spostate da un Ministero all'altro - lo abbiamo visto col PNRR - e poi trovate scuse, perché siete in ritardo sulle cose, allora tagliate e create problemi ai Comuni e alle Regioni, ma questi siete voi. *(Applausi)*. La passione incredibile per le *governance* vi ha portato a toccare anche quella a toccare anche quella del CSC, negandone, vincolandone o limitandone tantissimo l'autonomia e l'indipendenza e portando sotto il diretto controllo del Governo scelte e indirizzi riguanti percorsi che dovrebbero essere invece autonomi, perché riferiti alla docenza, agli strumenti formativi e alla didattica, che sono autonome per definizione: avete messo le mani quindi su un'istituzione culturale in un decreto della pubblica amministrazione, perché era quello che vi interessava. Nulla avete fatto invece per provare ad accelerare i problemi riscontrati sul PNRR e quindi dare più personale agli enti locali e alle pubbliche amministrazioni per lavorare meglio, ma d'altra parte lo avete certificato voi in Aula l'altro giorno con il ministro Musumeci, il quale è venuto a dirci che la media di tempo con cui si realizzano le opere in Italia sono cinque-sei anni a seconda dell'opera e per questo voi tagliate i progetti, dicendo che non faremo mai in tempo a realizzarli entro la scadenza del PNRR. Tuttavia, piuttosto che accelerare per fare in modo che questa media cambi, media cambi, non mettete un euro sul personale della pubblica amministrazione e così la situazione potrà solo peggiorare. Non solo non ci mettete un euro, ma spesso fate il gioco delle tre carte, perché i soldi li utilizzate solo per creare nuovi posti di diretta collaborazione per i Ministeri e andate a vedere. Signor Ministro, lei qui rappresenta tutto il Governo, ma le sembrano normali i nuovi posti che sono stati creati per le collaborazioni dirette dei Ministri? Le sembra una cosa sacrosanta in questo momento? *(Applausi)*. Noi che siamo per l'efficienza di un Governo e che riteniamo che sia giusto giusto che anche i Ministeri vengano messi nella condizione di lavorare, ci chiediamo come mai voi guardiate solo alla funzione e al lavoro del Ministro per le sue dirette collaborazioni, quindi scelte tutte sue e personali. Dicevo del gioco delle tre carte, che del gioco delle tre carte, che avete fatto rispetto al comparto scuola: si chiama decreto PA - e abbiamo detto che sta per personale apicale - ma direi che c'è una parte che riguarda la scuola rispetto alla quale non avete fatto nulla, se non ulteriori danni. del costo dei percorsi di abilitazione e di formazione iniziale degli studenti e di coloro che dovranno partecipare all'*iter* per

per aiutare i nostri ragazzi a diventare insegnanti. Il problema però è che dite a questi ragazzi di pagarsi da soli i corsi di formazione. Dite a questi ragazzi che vogliono diventare insegnanti che i costi devono gravare sulle loro famiglie e su di loro. Non mettete un euro neanche qui e, anzi, avete tolto gli euro, i soldi, che potevano servire per i percorsi abilitanti. Tra l'altro, trovo giustissimo che vengano integrati e migliorati gli incarichi del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). Il problema è che pagate questi incarichi con i soldi che erano stati destinati alla formazione dei nostri docenti. Vi rendete conto che non aggiungete i soldi per andare a colmare le lacune che ci sono, ma li togliete ad altri comparti? Onorevoli

dei nostri studenti. Avete detto di no anche al recupero dei tagli alla carta del docente. Con un nostro emendamento alla Camera dei deputati avevamo trovato le coperture, ma siccome rischiava di essere qualcosa a favore dell'opposizione, avete detto di no, meglio non farlo. Avete detto no ad un'altra cosa, secondo me davvero molto grave, perché non state favorendo la mobilità dei dirigenti scolastici che hanno vinto il concorso nel 2017,

di ottenere l'avvicinamento, perché quei posti sono stati messi a disposizione di altri. Non siamo contrari, ma vi chiediamo di trovare una modalità per consentire a quei dirigenti scolastici, che quel concorso lo hanno vinto subito e sono entrati in servizio, di avere dei canali Ministro, concludo con un'ultima battuta. Oggi, su un quotidiano, un autorevole esponente della maggioranza, noto ormai come il coinquilino, ha dichiarato che all'Italia serve un'opposizione seria e credibile. Credo però che al Paese serva un Governo serio e credibile un Esecutivo che usa due decreti per commissariare e sopprimere enti, consumare piccole vendette su vertici di istituti culturali, varare norme *ad personam*, togliere autonomia e indipendenza ad organi terzi e *super partes*, aumentare gli *staff* dei Ministeri e asservire al potere esecutivo i vertici apicali della pubblica amministrazione. Questo non si chiama buon governo, ma occupazione.

La Corte d'appello mi ha proclamata senatore. Non so a lei, collega: a me sì. PRESIDENTE. Chiamatevi come volete: senatrice o senatore, per me non è un problema. *(Applausi)*. Basta che lasciamo parlare il senatore Zedda. Onorevoli colleghi senatori, componenti del Governo, in questi mesi, ma in realtà da sempre, la sinistra ci ha portato spesso a una divisione: da una parte loro dall'altra tutti gli altri. Da una parte le categorie che dicono di difendere, come i lavoratori pubblici, i poveri, i buoni, i giusti e gli ultimi, mentre dall'altra ci siamo noi, i cattivi, i ladri, i lavoratori autonomi, gli omofobi, i razzisti, i credenti e gli oscurantisti. Poi si scopre la realtà: gli operai non votano più a sinistra da decenni a sinistra le donne che arrivano al potere le sceglie un gruppo ristretto di uomini, sino all'ultimo congresso, in cui una donna viene scelta da non tesserati del PD. I lavoratori dipendenti non ricevono migliorie della loro situazione, che voi giustamente raccontate, anche perché le conoscete bene. Ci sono tanti sindacalisti seduti fra come senatori e ci raccontano di situazioni di estremo disagio dei lavoratori dipendenti. Ma la sinistra cosa ha mai fatto per loro? Nelle periferie vince la destra. Nel centro di città quali Milano, Bologna - dove ha vinto sicuramente sempre la sinistra

Avete contrapposto fino all'eccesso il dipendente al lavoratore autonomo, alla partita IVA e all'imprenditore. Il indipendente ha uno stipendio basso, è vero, lo sappiamo tutti. Occorre agire: voi avete fatto qualcosa? No. Nuove assunzioni nel comparto pubblico, è vero, ce n'è bisogno: voi avete fatto qualcosa? No. Il dipendente non ha il rischio d'impresa, il suo datore di lavoro sì. Voi avete fatto qualcosa affinché il dipendente privato venga tutelato dal rischio d'impresa del suo datore di lavoro? No. Invece, dall'altra parte, ci sono i lavoratori autonomi e le partite IVA, che hanno il rischio d'impresa. Avete fatto qualcosa in questi anni per aiutare il libero professionista o l'imprenditore? No. Quante sono le partite IVA che hanno un lordo di 30.000 euro, ve lo siete mai chiesto? Secondo voi, queste partite IVA rendono ricchi? La risposta è no. Le avete mai aiutate? No. Sono evasori? No. E io sono tra quelli. Hanno le coperture per malattia e maternità, banalmente? La risposta è no. no. Questi primi nove mesi di Governo sembrano una gravidanza e la figlia che verrà fuori sarà una Patria forte, una Nazione credibile abbiamo ereditato una situazione drammatica e, oltre a tutto il resto, abbiamo avuto il tempo di emanare due decreti-legge per la pubblica amministrazione. È vero, dispiace non averli potuti analizzare con tempo e precisione al Senato, ma

è riservata agli *under* 30. Voi l'avete mai fatto? No. Opportunità per gli insegnanti, Forze dell'ordine, formazione dei dipendenti pubblici, potenziamento delle voi le avete mai considerate le ARPA? No. Incentivi per attrarre e trattenere ricercatori: cos'avete fatto voi, negli ultimi dieci anni? Noi non lo sappiamo, perché è un dato che non è pervenuto.

assolutamente, ma vi chiedo: ve ne siete accorti solo ora che noi siamo al Governo? Perché gli italiani se ne sono accorti da tempo e si vede, perché in maniera netta hanno fatto scelte elettorali non solo alle politiche, ma anche in tutte le Regioni. Non volete ascoltare un'altra affermazione: è un modo di governare che non può essere accettato. Ci avete lasciato un'eredità così pesante che o si corre o l'Italia muore, lo ripeterò all'infinito durante questa legislatura. confronto in sedi opportune, ad esempio le Commissioni, vorrei chiedere che venisse fatta un'analisi delle presenze, anche quando non sono previste votazioni, perché la maggioranza è sempre presente, la minoranza un po' meno. Attenzione a moltiplicare i posti dei dirigenti: abbiamo anche promosso assunzioni, come ho detto prima, non solo moltiplicato i dirigenti. Comprendo che a voi dia fastidio che si facciano selezioni senza di voi al Governo, ma così è la vita. Mentre voi avete fatto nomine discrezionali per anni e chiamate dirette, come ha detto anche la collega che mi ha preceduto, ad esempio per il Centro sperimentale di cinematografia, noi facciamo i bandi. Chi ha torto, le chiamate dirette o i bandi? *(Applausi)*. Comprendo vi diano fastidio tutta questa legalità, tutta questa meritocrazia e tutta questa trasparenza, ma sono l'unico modo che conosciamo per governare. Un SMS all'improvviso, ma davvero? A me non sembra, perché ci sono stati alcuni mesi di preparazione. Siamo pronti a dare dignità a tutti i cittadini italiani che altri hanno volutamente drogato. sistema carcerario, noi abbiamo assunto 30 dirigenti e più di 1.000 agenti; voi in cinque anni avete liberato i detenuti sottoposti al regime di 41-*bis* per Covid. Se aveste letto tutti gli articoli, avreste letto anche i numeri che voi non avete minimamente messo in moto in cinque anni. Colleghi, mi accingo a terminare non siamo saliti su nessun balcone e non lo faremo nemmeno oggi, perché abbiamo la coscienza che, pur avendo fatto tanto, ciò non sia quasi nulla per la situazione in cui versa l'Italia. Non abbiamo abolito la disoccupazione, la situazione di disagio in cui versa la pubblica amministrazione ci è nota e sappiamo che c'è ancora tanto da fare;

a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 829, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge legge 22 giugno

che la pubblica amministrazione è l'architrave dello Stato, è il fulcro attraverso il quale le istituzioni si relazionano con i cittadini e si occupano di soddisfare i bisogni della collettività e, secondo me, molta più considerazione anche presso l'opinione pubblica, che noi dovremmo accompagnare. Con questo provvedimento ampio e articolato, il Governo di centrodestra ha voluto continuare nell'opera di modernizzazione della macchina pubblica già inaugurata con il primo decreto-legge Esso infatti, al pari di altre iniziative legislative, segue un percorso per noi fondamentale: garantire una macchina pubblica e uno Stato più efficaci ed efficienti, secondo i *desiderata* del popolo italiano. Ciò perché crediamo che le famiglie italiane, le imprese e gli enti locali debbano avere una pubblica amministrazione elevata ad interfaccia tra lo Stato e cittadini, che non può essere invece ancora oggi un elemento che scoraggi e disincentivi, che renda l'utilizzo dei servizi pubblici che induca alla rinuncia chi abbia voglia di fare e di intraprendere. Il *mantra* di questo Governo di centrodestra è sburocratizzare. Al contrario, la pubblica amministrazione deve quindi essere una rete di sostegno e di protezione in grado di semplificare la vita ai cittadini e di avvicinare soprattutto le fasce più fragili e il mondo del lavoro e già oggi se ne sente il bisogno. Si tratta, signor Presidente, di una priorità assoluta e fin dal primo momento è stata interpretata come tale dal Governo di centrodestra e da questa maggioranza. La semplificazione delle procedure burocratiche è quindi un punto cruciale affrontato da questo decreto-legge, un obiettivo che avevamo scritto, come centrodestra, nel programma di legislatura e sul quale stiamo correndo, come ha detto prima una collega che mi ha preceduta, altrimenti, appunto, l'Italia muore, lo condivido pienamente. Ridurre la burocrazia significa ridurre gli ostacoli che spesso rallentano il processo decisionale e impediscono ai cittadini di accedere addirittura ai servizi pubblici. Semplificare le procedure significa rendere la pubblica amministrazione e quindi lo Stato - perché pubblica amministrazione e Stato si sovrappongono - più attraenti per gli investitori, promuovendo la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, perché la pubblica amministrazione dev'essere al servizio del cittadino e non viceversa, come purtroppo spesso accade. Nella nostra visione e in quella di questo Governo di centrodestra, c'è un'amministrazione pubblica snella, vicina ai cittadini e pronta ad ascoltare le esigenze e ad agire tempestivamente per soddisfarle. Questo decreto-legge mira dunque a ottimizzare le risorse umane e finanziarie della pubblica amministrazione: avere infatti una pubblica amministrazione efficiente non è solo un bene, ma ci permette di valorizzare

Paese più efficace, più snello e pronto alle nuove sfide, ha posto fine al reddito di cittadinanza *erga omnes* ed ha operato il taglio del cuneo fiscale, la semplificazione e l'agevolazione delle nuove assunzioni. Questi sono solo alcuni dei provvedimenti che, sommati anche al decreto-legge sul *made in* *Italy*, al provvedimento sul lavoro sportivo, alla tutela dei diritti d'autore e alla delega fiscale che abbiamo approvato ieri,

le radici cristiano-giudaiche nella nostra Costituzione). È quindi con la stessa motivazione che questo decreto-legge indica norme di programmazione e investimenti per la digitalizzazione dei cammini giubilari e del patrimonio sacro di Roma,

Ultimo, ma non meno importante aspetto che viene toccato dal decreto-legge è quello degli aiuti agli *asset* importanti del nostro Paese, cioè quelle aziende con un grande numero di dipendenti che potrebbero trovarsi in difficoltà, ma che noi abbiamo necessità che rimangano in Italia e magari che rimangano anche italiane, perché abbiamo già visto troppi *asset* italiani essere oggetto

voteremo quindi convintamente questo provvedimento, se non altro perché sia un chiaro esempio di come siamo pronti a intervenire, quando è necessario.

più trasparente e più capace di rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Noi crediamo che la modernizzazione della pubblica amministrazione sia

nonostante una serie di difficoltà che però sono emerse durante la fase di approvazione al Consiglio dei Ministri. In realtà, speravamo che il testo potesse essere corretto e adeguato dal Parlamento, tenendo conto anche delle esigenze reali del Paese, per provare ad offrire un segnale positivo alle pubbliche amministrazioni, che hanno bisogno di nuovo personale e di nuove competenze per rispondere alle richieste dei cittadini, ma purtroppo, dal nostro punto di vista, così non è stato. Abbiamo ascoltato quello che si è detto sulla scuola, sulla cultura, sulla difesa e sul tentativo, secondo me sbagliato, di ricostruire la *governance* dei Ministeri, senza valorizzare significativamente le personalità che pure all'interno dei Ministeri naturalmente ci sono e senza peraltro pensare al fatto che sarebbe stata necessaria una maggiore trasparenza. Ad esempio, a proposito del Ministero dell'istruzione e del merito, è stata inserita la possibilità di erogare i corsi abilitanti, praticamente tutti, con la cosiddetta modalità a distanza. Noi crediamo che questo sia stato fatto per andare incontro agli interessi delle università telematiche. Invece, siccome pensiamo che il successo della formazione non prescinda mai dalla relazione e dalla reciprocità tra chi insegna e chi apprende e che la modalità a distanza, in percentuale addirittura pari a quella in presenza, non sia utile agli aspiranti docenti, in molti casi anche privi di esperienza pregressa, crediamo che sia stato fatto un errore significativo, il contrario di quello che avevamo chiesto noi. noi. Questo provvedimento, naturalmente non soltanto per questa ragione, ma per un complesso di questioni, avrebbe quindi necessitato di essere migliorato,

questa sorta di difesa, per così dire, degli interessi particolari e questa forma di revanscismo, tra l'altro tipico delle vostre destre che governano il Paese, che pretende di cambiare tutto e di applicare norme che nella nostra Costituzione non ci sono, come ad esempio quella sullo *spoils system*. Ancora, il PNRR,

facendo fuoriuscire dal Piano le aree più a rischio. Come si è visto anche in occasione dell'ultima drammatica alluvione dell'Emilia Romagna, pur avendo detto che avreste messo tutto a posto e avreste dato un segnale a quel territorio,

dal nostro punto di vista particolarmente significativi. L'abbiamo già detto in altre occasioni: tagliate i fondi per mettere in sicurezza i fiumi del Paese, mettete in discussione i soldi per avviare

per funzionare (quindi anche i funzionari e i dipendenti). Gli organici dei Comuni - lo sappiamo e lo sanno tutti coloro che negli anni hanno avuto a che fare con gli enti locali - sono ridotti all'osso, ma voi continuate a tagliare e continuate a insistere su questo. In realtà, in questo modo tagliate i bisogni e i servizi dei cittadini e peraltro lo fate esattamente in contemporanea - ne discuteremo oggi pomeriggio - all'operazione davvero scellerata che avete fatto in queste ore. Veramente la definisco una delle più grandi operazioni di crudeltà sociale fatta negli ultimi anni *(Applausi)*: lo scellerato SMS con il quale avete comunicato a 169.000 cittadini *(Applausi)* che non avranno più un reddito.

come sappiamo bene - sono sopravvissute in questi anni grazie al reddito di cittadinanza; persone che inevitabilmente andranno dai loro sindaci a chiedere un aiuto e andranno a rivolgersi ad amministrazioni comunali che però non sanno nemmeno bene cosa rispondere, perché le loro finanze sono ridotte all'osso e anche i programmi del PNRR sono stati significativamente cambiati. Francamente, credo che questo inaccettabile scaricabile che state facendo sui Comuni sia davvero così esemplare del fatto - mi dispiace dirlo, ma è così - che non avete più niente di quella destra sociale che avete sbandierato durante la campagna elettorale. Siete una destra liberista, ultraliberista, in totale continuità - da questo punto di vista - con trent'anni di politiche economiche liberiste, e davvero mi dispiace molto che abbiate abbandonato alla propaganda elettorale quegli elementi e quei risvolti sociali che invece pure avevate sbandierato, ma che evidentemente sono rimasti lettera morta. Questa purtroppo è la realtà.

tutte le funzioni del Comitato per la previdenza complementare ad Assoprevidenza, che è una struttura privata, con 29,5 milioni di euro di finanziamenti pubblici. Anche il fatto che si scelga di procedere in questo modo, senza coinvolgere al tavolo il Ministero del lavoro, mi pare francamente molto, molto discutibile. Davvero non mi è chiaro quando si farà in modo che a quei lavoratori e a quelle lavoratrici del pubblico impiego venga riconosciuta la dignità, vengano riconosciuti anche quegli aumenti necessari per poter svolgere il loro lavoro; quando verranno indetti i pubblici concorsi per reclutare una nuova generazione di dirigenti nei Comuni, per promuovere quel rinnovamento generazionale che invece servirebbe moltissimo. Lo sappiamo: l'età media dei dipendenti pubblici è molto elevata, ma su tali questioni non ci sono accenni nel vostro decreto-legge. Avete discusso di una serie di tematiche, ma avete ignorato questi punti cruciali. Da questo punto di vista, credo davvero che occorrerebbe una svolta, che però non si vede. Sarebbe necessario ottenere una pubblica amministrazione efficiente e di alta qualità; servirebbe un salto di qualità significativo. Avreste probabilmente dovuto accettare anche un vero confronto con le opposizioni e con le parti sociali, che hanno contestato questi provvedimenti su quei problemi concreti che riguardano la vita quotidiana di ciascuno di noi e, in particolare, il futuro delle giovani generazioni che oggi frequentano le scuole. scuole. Crediamo che sarebbe servito un dibattito serio su questi grandi nodi aperti del Paese. Invece, purtroppo, ci sembra che abbiate perso un'altra opportunità

che andando avanti in questo modo la condizione sociale del Paese peggiorerà ancora di più. Mi dispiace molto, ma è l'ennesima occasione perduta. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, abbiamo il secondo decreto-legge per la PA dopo poche settimane dall'approvazione del primo

Una pubblica amministrazione efficace e preparata è quella che ci fa portare a casa il PNRR trasversalmente. Abbiamo visto in questi mesi,

un blocco importante. Per questo credo che dalle pagine dei giornali un presidente che non appartiene al mio Gruppo politico come Fedriga, che in questo momento rappresenta le Regioni, gridi

amministrazione. Posto che io credo, come il suo predecessore, il ministro Brunetta, che la riforma Bassanini debba essere modificata, attuata e attualizzata perché sono passati decenni. Oggi possiamo fare un tagliando di quello che ha funzionato e di quello che non ha funzionato, senza nostalgie e senza dire che, quando la sinistra ha governato, ha fatto solo danni perché quel provvedimento nacque, per esempio, da una risposta sulla macchina pubblica contro la corruzione. È stato uno degli effetti di Tangentopoli prevedere una ripartizione diversa tra potere politico e potere amministrativo. Oggi però possiamo dire che la paura della firma blocca due terzi delle autorizzazioni e i nostri imprenditori nostri ci chiedono semplicità proprio per questo *(Applausi)*, perché è più facile fare impresa all'estero, ad esempio, in Paesi come la Francia, dove non si può dire che lo Stato centrale non sia forte o lo Stato periferico attuale, o la Germania, dove abbiamo uno Stato federale che è ancora più forte dello Stato centrale. Eppure l'Italia - non so perché - non vuole essere semplice. Questo provvedimento serve - beati loro promuovere alcune persone in alcuni Ministeri. Io non ho mai invidia sociale; tutti meritano di essere accontentati e beati loro, buon lavoro e buona fortuna e speriamo che ci diano una mano per il nostro Paese. *(Applausi)*. ai dipendenti pubblici, non fa la selezione di merito che servirebbe. Secondo me in questi anni abbiamo anche raccontato male la pubblica amministrazione. le persone che vanno a lavorare nel pubblico impiego più o meno si facciano la *manicure* dalle 8 del mattino alle 17 e poi se ne vanno via, e invece no. Se questo Paese, è di eroi non è soltanto perché abbiamo le imprese con imprenditori lungimiranti, ma anche perché abbiamo dei lavoratori che si assumono le proprie responsabilità *(Applausi)*, anche se non vengono premiati. Un'altra cosa che infatti non c'è è il premio per chi fa. Se vogliamo incentivare la mancanza di paura di firma, oltre a quello che prevede la riforma Nordio - è per quello che noi ne parliamo positivamente: togliere l'abuso d'ufficio non è una questione da poco sul terrore alla firma

Anche sulla formazione, mi aspettavo una continuità rispetto al suo predecessore Renato Brunetta che, con la ministra Messa, fece un accordo per incentivare le lauree dei pubblici funzionari, funzionari, centrando un obiettivo del PNRR, il punto 1.1, nel quale si dice che la pubblica amministrazione incentiva anche economicamente la possibilità di frequentare università e master, che tendenzialmente sono molto costosi, per cui non tutti possono permetterseli. Lei ha fatto accordi con tre università telematiche - beate loro - ma, secondo l'ANVUR, non hanno le caratteristiche per fare le stesse cose delle università in presenza sul modello Brunetta. Oggi con il decreto in esame questo anche alla formazione degli insegnanti. E meno male che sono stati cancellati gli emendamenti che non prevedevano la presenza in video e la possibilità di registrare la lezione e sbobinarla a tempo debito.

il Covid. Gli obiettivi del PNRR sono di riprendere un Paese che ha avuto la più grande tragedia a causa del Covid, non soltanto per le morti ovviamente, ma perché non era pronto a superare un'emergenza così drammatica. Invece, stiamo sprecando delle risorse per degli incentivi *ad personam* e non per fare della pubblica amministrazione una macchina efficiente ed efficace. I tempi di attesa che ogni persona ha rispetto a una burocrazia che gli è nemica fanno sì che il cittadino abbia sfiducia nei confronti dello Stato.

non ci sono dipendenti nei grandi Comuni, figuriamoci nei piccoli. Vorrà dire che la sarà la classe politica, il sindaco di turno di un piccolo paese, a doversi prendere la responsabilità di dare risposte ai cittadini infuriati senza avere le prebende dei parlamentari, con buona pace di chi si lamenta dei nostri stipendi. Forse allora è arrivato il momento di sederci tutti attorno a un tavolo, maggioranza e opposizione, per dire che cosa vogliamo fare del Paese. Quali sono le tre riforme importanti da qui a fine legislatura che ci possono dare una mano per raggiungere i risultati del PNRR? Perdere un solo euro di quelle risorse vuol dire danneggiare il Paese tre volte: dire all'Europa che noi non siamo in grado di spendere i soldi europei; dire agli italiani che non abbiamo capito niente dall'emergenza e, soprattutto, non dare la possibilità a questo Paese di rinascere definitivamente in modo serio. Allora, signor Ministro, signor Presidente, noi voteremo contro la fiducia e contro questo provvedimento, anche se non ci fosse stata la fiducia, perché è un provvedimento non sulla pubblica amministrazione, ma per alcuni fortunati che - beati loro - avranno la possibilità di essere assunti in qualche Ministero. Con questo provvedimento non si cambia assolutamente la realtà della pubblica amministrazione e non si dà neanche una visione d'insieme su dove si deve andare. Il PNRR individua compiti specifici e delle missioni incredibili su tutti gli argomenti e, in particolare, su questo. Mi auguro che nelle prossime puntate, perché ci sarà un decreto PA 3 - tipo Rocky, Rocky 1 con Adriana sconfitto, interpreterà - i protagonisti siano la pubblica amministrazione, i dipendenti e la capacità di renderla più snella.

di assunzioni - dirigenziali e non - e delle proroghe di incarichi: ciò è necessario al funzionamento dei dipartimenti interessati, con particolare rilievo anche per tutti gli interventi relativi al PNRR. Cito alcune delle tante disposizioni, cominciando da quella per garantire la piena operatività delle reti oncologiche regionali, con il parere delle associazioni dei malati oncologici e con precisi indicatori a livello nazionale in tutte le Regioni. Su questo tema - ahimè - ho una particolare sensibilità. Sono previste misure di semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure di contrasto del cosiddetto rincaro dei materiali. Viene differito dal 15 gennaio 2024 il termine per rendere operativa la cosiddetta riforma Cartabia del processo penale. Si provvede anche a modificare la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e di abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie. Sono previste anche disposizioni in materia di formazione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno. Per quanto riguarda la mia Sicilia, viene disciplinata la gestione del fondo per il sostegno dei Comuni in *deficit* strutturale, che consentirà la ripartizione delle risorse anche ai Comuni nelle Regioni Sicilia e Sardegna, che prima erano state erano state escluse in quanto a Statuto speciale. In materia di agricoltura, vengono assegnate ulteriori risorse per interventi a sostegno delle aziende agricole e per aggiornare i vari sistemi di controllo di AGEA che danno informazioni per il comparto zootecnico. Per quanto riguarda lo sport, è prevista una serie di interventi volti alla semplificazione delle attività per l'organizzazione dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 inoltre si prevede anche una serie di agevolazioni e adeguamenti statuari per tutte le società aderenti al CONI e alle varie federazioni sportive nazionali ad esso associate. Infine, si autorizza la spesa per la Santa Sede per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. Riteniamo che il decreto-legge preveda una serie di disposizioni per rendere più funzionale la pubblica amministrazione.

Presidente, vorrei partire da una considerazione preliminare. Ci siamo resi conto che abbiamo a che fare con un provvedimento multidisciplinare, un insieme eterogeneo di norme che non si sa come sono legate insieme; una sorta di macedonia normativa che qualche problema ce lo deve porre. C'è dentro un po' di tutto, dall'agricoltura allo sport, dal lavoro al Giubileo. All'interno di queste macro-categorie ci sono tante altre sotto-categorie e, quindi, si parla anche dei magistrati onorari o dell'Agenzia italiana del farmaco. Ci sono tantissime misure, ma tante altre sono rimaste fuori e non a caso. Purtroppo sono rimaste fuori perché ancora una volta si è fatta la scelta della decretazione d'urgenza.

Fatemi capire: anche se ce ne fosse uno di provvedimento urgente, tutti gli altri cosa c'entrano? Perché dovete sottrarvi al normale dialogo parlamentare? A me sembra che non ci sia nulla di urgente, ma non esiste una *vis* attrattiva che vi consente di mettere dentro un po' di tutto e scavalcare le regole normali e ordinarie. e ordinarie. Ripeto ancora una volta la domanda, ma questa volta ritengo che sia ancora più doveroso da parte vostra darci delle risposte. Se tutto diventa urgente - come sta dimostrando il Governo con l'ennesima

Presidente, colleghi di maggioranza, non è un problema legato soltanto al rispetto delle regole democratiche. È un problema di rispetto della nostra Costituzione, di rispetto dei cittadini che anche noi di opposizione vogliamo rappresentare. Non potete interrompere il dialogo democratico. Non potete fare un provvedimento che lascia fuori troppi argomenti perché non c'è tempo di affrontarli, perché abbiamo tempi stretti legati al bisogno di convertire un decreto-legge e questo non consente un sano dialogo democratico. È significativo che anche il Capo dello Stato abbia rivolto un invito a dare valore al dialogo parlamentare. Si parla di dibattito parlamentare in Aula, Aula, il dialogo democratico. Questo è il senso vero della democrazia: il rispetto che si deve avere nei confronti della popolazione che rappresentiamo. Stavo facendo una riflessione sul progetto politico di insieme. Mi sembra che, oltre al fatto che a volte si fanno provvedimenti frettolosi come questo,

Ma o i problemi non li si risolve o addirittura se ne creano più di quanti non se ne vogliano immaginare di risolvere. Facciamo un altro esempio: in Italia abbiamo un livello crescente di disoccupazione. intere aree territoriali - parlo non solo di quelle delle Regioni del Sud, ma anche delle aree di crisi industriale complessa - dove bisogna creare sviluppo e occupazione; bisogna investire e creare posti di lavoro. Ma il Governo che cosa sta facendo? Elimina il reddito di cittadinanza.

Ve ne posso presentare migliaia di occupabili del mio territorio. Ce ne sono tanti di occupabili, ma abbiamo una zona industriale dove dove il 50 per cento delle aziende ha chiuso. Mi sa dire dove possiamo collocare quelle persone che non hanno lavoro? L'unica possibilità è creare sviluppo, investire, ma a quanto pare gli investimenti vanno un po' a monte, visto che quasi 16 miliardi del PNRR non vengono più investiti. *(Applausi)*. Spariscono miliardi per le infrastrutture, miliardi per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Stiamo facendo l'esatto contrario di quello che non solo il buon senso suggerisce, ma di quello che hanno capito altri Paesi europei. Andate a vedere cosa ha fatto la Spagna, che investe nello sviluppo delle infrastrutture e incentiva la creazione di posti di lavoro. Guardate l'Irlanda, guardate la Germania. Non sono nuove queste politiche di sviluppo: la Germania, già quando è caduto il muro di Berlino, ha immediatamente messo in atto politiche di sviluppo per evitare i divari territoriali. Noi che cosa facciamo, invece? Cerchiamo di creare nelle Regioni più povere una *bad company*, una *bad company*, mettendo in campo un modello, quello dell'autonomia differenziata, che può funzionare in Germania dove non ci sono divergenze territoriali, ma in Italia è come mettere un paio di scarpe strette con le quali non si riesce a camminare. Ancora, dobbiamo affrontare il problema delle Province. Chiedete a qualunque cittadino: qual è il problema delle Province? Non ci sono i soldi per fare le strade;

perché non ci sono i soldi. Quindi, se si fa una riforma delle Province, Presidente, io penso che bisognerebbe mettere in campo un sistema che vada a finanziare e dare i soldi alle Province per mettere a posto le strade. La prima cosa che si fa, invece, è cambiare i criteri di nomina dei presidenti e andare a creare nuove poltrone. Ecco, su questo il MoVimento 5 Stelle non ci sta.

alle quali il MoVimento ha cercato di rimediare. Già alla Camera i colleghi hanno presentato degli ordini del giorno per cercare di migliorare un provvedimento che poteva essere sicuramente migliorato, nel quale c'erano molti spazi. Tutti gli emendamenti, però, del MoVimento 5 Stelle sono stati bocciati; per fortuna qualche ordine del giorno è stato accolto, impegnando il Governo, ad allineare le retribuzioni dei vigili del fuoco durante gli orari notturni e festivi con quelle delle Forze di polizia. Sono piccole cose che vengono fatte perché il MoVimento 5 Stelle sta vicino ai cittadini, applica una politica partecipativa, vuole ascoltare. Come facciamo a dare ascolto alla popolazione se poi c'è la tagliola perché non si possono più fare emendamenti? Qui al Senato non possiamo fare nulla

Quando non si ascoltano le opposizioni, significa non ascoltare le istanze che arrivano da una parte importante della popolazione. Desidero quindi invitare la maggioranza a una grande riflessione su questo punto: cerchiamo di pensare di fare una politica nuova. Peraltro, la scelta della decretazione d'urgenza è uno dei problemi tipizzanti dell'Italia. Se provate a confrontarvi con i parlamentari di altri Paesi europei, scoprirete che l'Italia ha questo fiore all'occhiello

amministrazioni centrali. È inutile che vi ricordi che non ho competenze specifiche per tutti gli argomenti trattati, ma per i temi che conosco discretamente consentitemi, per rafforzare il concetto della necessità del decreto-legge in votazione, di soffermarmi sulla parte sanitaria, sia umana che animale e agroalimentare, considerato che da essa discende lo stato di salute e benessere dell'intera popolazione.

Non che il problema sia nato un mese fa: il problema è noto almeno da un decennio, ma il decreto-legge in esame finalmente pone le condizioni per finalizzare le risorse incrementali specifiche già stanziate e per ottimizzare le reti oncologiche regionali e il coordinamento generale, a garanzia di piena operatività in tutto il Paese e con la messa a regime dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza, grazie anche al referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. strumenti e meccanismi normativi di immediata applicazione in forza di decreto, che consentiranno di fare prevenzione vera e dunque di favorire l'implementazione attualizzata - in ragione di quanto già fatto suo dal Governo - degli ordinamentali, che sono in avanzata fase di elaborazione. Mai infatti come in questo periodo, consapevoli della centralità della salute anche per lo sviluppo economico, dobbiamo lavorare a un miglioramento continuo dell'accessibilità, della qualità e dell'equità delle cure, soprattutto in emergenza-urgenza e assistenza territoriale, puntando sul coinvolgimento proattivo dei medici del ruolo unico di assistenza primaria, non solo negli *screening* oncologici consolidati, ma anche in evoluti programmi di prevenzione e promozione della salute, da cui muove la lotta ai tumori. ciò incontrerebbe serie difficoltà in assenza di quanto previsto dal decreto-legge in conversione. Agendo in prevenzione primaria, secondaria e terziaria sui fattori di rischio prevedibili e la diagnosi precoce, si recupererebbero quindi non solo i ritardi diagnostici, ma si raggiungerebbero anche i livelli di copertura ottimali dei programmi di *screening* superando le disparità territoriali. Prevenzione e controlli sistematizzati per dare di più anche in innovazioni farmacologiche e terapie avanzate, rafforzando quantitativamente e qualitativamente Aifa, per una rapido esame dei *dossier*, soprattutto quelli relativi alle terapie innovative. Questo è lo spirito con cui il decreto-legge n. 75 che andiamo a convertire si prospetta, ponendo rimedio con immediati benefici alle più urgenti necessità di tutta la filiera del sistema Paese. Credetemi: di sanità sono trent'anni che me ne occupo e dei contenuti di questo provvedimento c'era bisogno, in particolare per la diagnosi precoce e la medicina predittiva, dove abbiamo previsto che potranno essere finalizzate maggiori risorse come già suggerito in occasione della discussione della legge di bilancio - finalizzate a testi genomici che eviteranno fino all'80 per cento la chemioterapia, con l'innalzamento della qualità della vita dei pazienti e il contenimento dei costi indotti. Ma senza dei registri tumori generali e specializzati integrati, alimentati correttamente e in continuo si possono fare in buona fede errori sesquipedali nella programmazione. Sono all'esame della 10a Commissione due disegni di legge, il n. 224 e il n. 227, a cui stiamo lavorando da tempo con lo scopo di rafforzare la medicina territoriale per risposte immediate ai bisogni che non richiedono ospedalizzazione, intervenendo normativamente con un modello di continuità nell'assistenza e cura basato sul rilancio del medico di medicina generale e per un riordino dell'emergenza-urgenza di effettiva continuità assistenziale ospedale-territorio che dia certezza di di appropriata e tempestiva presa in carico delle patologie tempo-dipendenti, sgravando per un verso i pronti soccorso dal carico della domanda che non richiede ospedalizzazione, per altro verso liberando risorse umane e strumentali per diagnostica preventiva, prestazioni e degenze per l'elezione, attività di approfondimento e di intervento specialistico ad elevata complessità e intensità di cura, precondizioni di fattibilità per la normalizzazione delle liste d'attesa. Ma senza quanto dedotto nel decreto in conversione tutto quanto prospettato come passo successivo sarebbe di più difficile implementazione, con ciò essendo quasi certi di contrastare l'utilizzo inappropriato dei pronti soccorso per un buon 25-30 per cento, nel quadro di un'integrazione dell'emergenza-urgenza preospedaliera e ospedaliera che affronta le debolezze e criticità di sistema sia sul piano del necessario investimento in capitale umano che in innovazione non solo tecnologica, ma organizzativa e funzionale, razionalizzando inefficienze e disfunzioni grazie ad un sistema di valutazione delle *performance* ispirato alla prevenzione e all'appropriatezza, dando voce all'esperienza delle associazioni. Efficientando l'intera filiera medicina territoriale-emergenza-urgenza, con effettiva digitalizzazione di quelli che sono i processi per sburocratizzare e tracciare, riteniamo si vadano a riorientare

ai necessari processi di riordino. Anche in questo senso, il rafforzamento delle strutture ministeriali sarà di supporto alla completa attuazione, a controprova che il vero tema è la corretta e appropriata finalizzazione delle risorse disponibili, con effetto moltiplicatore e generatore di valore, attraverso la tracciabilità degli impieghi e il controllo degli esiti, in ossequio al basilare principio "dove li prendo, dove li metto, cosa ne faccio". Da qui la necessità di una forte *governance* pubblica nella prevenzione, programmazione e acquisto, con sistema di valutazione, monitoraggio e controllo di tutti gli erogatori secondo flussi amministrativi parlanti, vale a dire dati e informazioni opportunamente calibrati per l'analisi, la valutazione e il controllo istituzionale, incentivando le pratiche virtuose e remunerando adeguatamente prevenzione e appropriatezza, anche per quanto riguarda tutta la filiera dell'agroalimentare. Così l'articolo 29 per la prevenzione e il contrasto della peste suina, incidendo nella gestione commissariale per la sua eradicazione, e l'articolo 30 per il potenziamento dei controlli degli agroalimenti e di contrasto alle frodi. Anche in questa prospettiva, peraltro, con l'ordinamentale n. 225, si andrà a completare il tutto, in modo tale da garantire il rafforzamento della sanità veterinaria e della sicurezza alimentare, con un sistema globale di valutazione del benessere del consumatore, mediante integrazione con la filiera agroalimentare e la qualità del benessere animale, in una visione normativa tesa a far scuola per le direttive europee, atteso che - come ho già avuto modo di dire - il tutto deve essere proiettabile in una dimensione applicativa sovranazionale, capace di far incrementare il nostro *market share* verso quei mercati molto attenti alla qualità e ai controlli degli agroalimenti. Quindi, come del pari non mi stancherò mai di sottolineare, in una prismatica strategia di cultura della prevenzione, che è alla base della sanità del futuro, iniziando il vero cambiamento. A questo punto potremmo immaginare di ammodernare l'intera filiera, andando normativamente a sostenere e debitamente a suggerire al mondo agroindustriale delle innovazioni in approccio *one-health*, a salvaguardia della salute di tutti, che per esempio permettano, mediante controlli da remoto, di utilizzare molti meno antibiotici di quanti non ne vengano attualmente impiegati; di usare meno acqua di quanta attualmente se ne sprechi; in una sola parola, proiettare il nostro Paese nel futuro, dotandolo di infrastrutture che ne cambino radicalmente il modo di concepire la tradizione con l'innovazione, promuovendo le vere eccellenze del *made in Italy* e i sani stili di vita che preservano la salute dei consumatori. Tutto quanto contenuto nel decreto-legge n. 75 va in questa direzione. Le ragioni, che in via meramente esemplificativa vi ho espresso, sono infatti *de plano* immediatamente e circostanziatamente estensibili alle restanti disposizioni in decretazione e, per ciò stesso,

Presidente, noi siamo in preda a un sentimento di rammarico e di delusione, perché ritenevamo che in materia di pubblica amministrazione fosse necessario un provvedimento audace e ben fatto. Invece, ci ritroviamo di fronte all'ennesimo provvedimento modesto e sbagliato. Prima ancora di qualsiasi considerazione di merito - del resto ne hanno fatte molte i colleghi che per il mio Gruppo e per gli altri Gruppi di opposizione sono intervenuti in questo dibattito - vorrei però fare una considerazione di metodo, che ha a che fare con la protratta e sempre più grave umiliazione del Parlamento a cui stiamo assistendo un ricorso ormai spasmodico da parte del Governo alla decretazione d'urgenza, seguita dall'apposizione di questioni di fiducia e di voti di fiducia. Quando si sono svolte le elezioni, abbiamo sentito la maggioranza dichiarare con molta forza che si apriva una fase nuova, perché c'era un mandato elettorale chiaro a una coalizione che aveva vinto le elezioni; questa coalizione aveva raccolto il 60 per cento dei seggi e sarebbe stato perciò possibile seguire le vie ordinarie in Parlamento e consentire al Parlamento di esprimersi sui provvedimenti, perché numeri così larghi avrebbero finalmente creato un'epoca in cui il ricorso ai decreti sarebbe stato residuale e ridotto. Questo film non è andato in onda, o è andato in onda su schermi che non sono nella nostra disponibilità. I numeri sono infatti effettivamente larghi, ma ancora più largo è il ricorso alla decretazione d'urgenza che comprime la possibilità del Parlamento di svolgere il proprio ruolo. Questo problema non dovrebbe sentirlo come grave soltanto la minoranza, ma dovrebbe sentirlo come grave anche la maggioranza, che dovrebbe avvertire che c'è una lesione della dignità e delle prerogative del Parlamento e prendere le dovute contromisure. Questo non sta avvenendo. In materia di pubblica amministrazione, siamo di fronte oggi alla necessità di dare una valutazione sul che è stato emanato il 21 giugno, promulgato in quella data, entrato in vigore il giorno successivo e frettolosamente esaminato alla Camera. È arrivato al Senato completamente inemendabile e inesaminabile, ma soltanto giudicabile - come stiamo facendo oggi - in sede di dibattito finale in Aula, dove ognuno di noi dice se è favorevole o contrario (noi ovviamente siamo contrari), ma senza aver avuto la minima possibilità di incidere sul merito del provvedimento. Tale procedimento richiama nel titolo l'organizzazione della pubblica amministrazione e mi viene da fare questa considerazione: PA, che l'Assemblea del Senato ha votato definitivamente il 20 giugno, quindi poche settimane fa, recava nel titolo l'obiettivo del miglioramento delle capacità amministrative della pubblica amministrazione. Ora la maggioranza mi pare sia in rapida discesa sul livello delle ambizioni: il miglioramento delle capacità della pubblica amministrazione scompare anche dai titoli dei provvedimenti; ci si limita all'organizzazione, però purtroppo mi pare che la qualità delle scelte che si fanno sia in costante peggioramento. I colleghi intervenuti prima di me hanno sottolineato bene le tante cose che non vanno in questo provvedimento. Io non voglio fare un elenco lungo e mi concentrerò

e che sarebbe adeguato al merito delle scelte che sono state compiute. Le porcherie riguardano un emendamento inserito nottetempo alla Camera. Apro e chiudo una parentesi: il provvedimento è arrivato alla Camera con 45 articoli e ne è uscito con 76, quindi già non poter esaminare un decreto-legge in un'Aula del Parlamento è grave; ma non poter esaminare un decreto che nell'altra Camera è quasi raddoppiato è doppiamente grave. La prima porcheria, come dicevo, riguarda un emendamento che mi risulta essere stato proposto e approvato nottetempo dalla Camera, che sostanzialmente fa uno scippo sulla previdenza complementare, perché sottrae al Comitato per la previdenza complementare una competenza e l'affida all'associazione Assoprevidenza, con uno schiaffo inutile ma molto grave alle parti sociali, le quali vengono private di qualsiasi ruolo in una materia decisiva senza che ci sia stata nessuna informazione preventiva e nessun confronto preventivo. Ma che modo di fare è questo? Stiamo parlando della previdenza complementare; stiamo parlando di una cosa che, come sappiamo tutti dalle ultime riforme previdenziali, è decisiva per il potere d'acquisto futuro dei pensionati a più basso reddito. Come mai non vi viene mai in mente di porvi il problema di che cosa serve, di che cosa è più utile per le classi di reddito di questo Paese, che sono medie e basse? Come potete pensare che la confluenza del Comitato per la previdenza complementare in Assoprevidenza possa essere una misura utile, giusta e comprensibile? Noi abbiamo presentato un emendamento soppressivo a questa misura, ma ovviamente - ripeto - il contesto in cui l'abbiamo fatto è quello di una discussione che è pure accademia, perché il Senato non può emendare, non può esaminare, non può dire niente: può soltanto scegliere se timbrare o non timbrare sotto il ricatto di una scadenza più o meno imminente. Quindi questa porcheria la possiamo denunciare e lo stiamo facendo; è una porcheria molto grave. Che dire dell'altra porcheria che mi sento di segnalare in sede di dichiarazione di voto? È quella che riguarda il colpo di mano che è stato attuato - non so se nottetempo oppure no, ma poco importa il periodo della giornata in cui è avvenuto - contro la fondazione Centro sperimentale di cinematografia contro la quale è stato applicato il sistema già sperimentato per INAIL e per INPS del commissariamento propedeutico all'occupazione. Il titolo giusto dei provvedimenti che state facendo, sia del decreto-legge cosiddetto PA 1 che del decreto-legge PA 2, non dovrebbe riguardare il miglioramento o la modernizzazione della pubblica amministrazione. Il titolo dovrebbe essere: misure urgenti per la lottizzazione interna alla maggioranza della pubblica amministrazione. è l'unico scopo che viene perseguito con coerenza e con vigore in questi provvedimenti che, in così rapida successione, sono stati presentati all'esame e al voto del Parlamento. Di tutte le cose che si possono fare come colpo di mano, come *blitz*, come cosa davvero di basso livello, quelle che si compiono contro la libertà e l'indipendenza della cultura sono tra le più gravi. *(Applausi)*. La porcheria fatta contro il Centro sperimentale di cinematografia è un attentato alla libertà e all'indipendenza della cultura, risponde soltanto a una voglia famelica di mettere le mani su tutto quello che si pensa si pensa possa produrre una qualche rendita in termini di potere e di controllo sociale. Tutto questo però è molto sbagliato. Vengo rapidamente, per concludere, alle due grosse lacune che corrispondono a un danno che si fa a tutto il Paese. noi siamo stati messi di fronte in questi ultimi giorni a un'azione, che per la maggioranza dovrebbe essere avvilente e che dal nostro punto di vista è nauseante: la guerra la guerra ai poveri attraverso il taglio di parte importante degli assegni del reddito di cittadinanza che vengono corrisposti nel nostro Paese. Ora, mentre si fa un'azione del genere si potrebbe, anzi si sarebbe dovuta sentire la necessità di affiancare a un'azione che comunque noi non condividiamo, un investimento perlomeno di carattere eccezionale per favorire il reinserimento lavorativo, l'occupabilità e quindi l'esigenza di mettere in campo un grande Piano nazionale per la formazione e per la riqualificazione professionale. Tutto questo è stato fatto? No, PA, che riguarda l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e nemmeno più si pone il problema di migliorare la capacità amministrativa delle stesse, si introduce la soppressione dell'ANPAL che viene soppressa e sostituita da che cosa? Da niente. Lo Stato dichiara cioè di essere impotente sulla formazione professionale, il Governo dichiara di non avere uno straccio di idea su come si possono incrociare meglio domanda e offerta di lavoro, su come si possono dotare le persone delle competenze necessarie per inserirsi bene nel mondo del lavoro o per reinserirsi, se ne sono uscite, su come si migliora l'occupabilità, su come si fanno investimenti sul capitale umano. Non c'è uno straccio di idea. Si sopprime l'ente che dovrebbe perseguire questi scopi, si richiamano le competenze all'interno del Ministero del lavoro, dove questi questi tentativi finiranno sepolti da non si sa che cosa e certamente produrranno il niente. È una cosa molto grave per l'Italia. La seconda cosa altrettanto grave è è che stiamo discutendo ormai da settimane dei pasticci, dei fallimenti, delle zoppie, che l'attuazione del PNRR in Italia sta conoscendo per vostro demerito. Ora, in una fase come questa, in cui avete seminato angoscia e preoccupazione negli enti locali e nelle Regioni, che ovviamente vedono a rischio investimenti importanti, non sanno se cose che hanno legittimamente affidato, appaltato e in qualche caso contrattualizzato, potranno arrivare a termine perché c'è una promessa vaga di fondi che però non sono stati stanziati e non si sa precisamente da dove verranno. Siamo alle assicurazioni più che generiche, alle assicurazioni metafisiche; queste sono le assicurazioni del ministro Fitto. A queste pubbliche amministrazioni si poteva dare con questo provvedimento il messaggio che, nonostante queste incertezze, nonostante questa nube di incompetenza che avvolge l'attuazione del PNRR, perlomeno si considerava il potenziamento vero, la modernizzazione vera della pubblica amministrazione, un grande obiettivo del Governo e del Paese. Ma non è affatto questo che anima il L'obiettivo della modernizzazione e del potenziamento della pubblica amministrazione in questo Paese non ve lo siete proprio posti, nemmeno per sbaglio. *(Applausi)*. Niente sulla scuola. Niente sulla sanità. Niente sulla stabilizzazione dei precari al Ministero della giustizia per l'ufficio del processo. Questo provvedimento ha soltanto un grande obiettivo: moltiplicare la spesa per le posizioni apicali, fare infornate di posizioni e di *staff*, proseguire quella lottizzazione interna alla maggioranza di cui parlavo prima. Per il personale comune della PA, cioè per quelle persone, quelle donne e quegli uomini, da cui dipende davvero la capacità della PA di portare a termine i propri compiti, c'è soltanto una grande disattenzione

e delle ambizioni con cui vi presenterete di fronte al Paese continuerà inesorabilmente. Per tutte queste ragioni siamo contrari al provvedimento, contrari alla fiducia ed estremamente preoccupati per come vi state comportando.

un'azione concreta attraverso la quale si sta costruendo l'Italia del futuro, una Nazione moderna, competitiva, attrattiva. Una Nazione che cresce e che vuole continuare a farlo con un serio rinnovamento, capace di portare alla realizzazione di un ambizioso progetto di riforme per adeguare la nostra pubblica amministrazione e renderla capace di dare finalmente risposte giuste ed efficaci alle esigenze dei cittadini e, soprattutto, di essere all'altezza, in termini di operatività ed efficienza, di attuare un piano straordinario come il PNRR, che prevede complesse procedure di gestione per l'ammodernamento del Paese. Presidente, si è detto fino ad ora che questo provvedimento è modesto, sbagliato inefficace. Ma di cosa stiamo parlando?

per rispondere solo alla politica della *spending review*, un *turnover* che non è mai iniziato, quando, se una sola persona manca nei piccoli Comuni, diventa veramente una tragedia. Ma di che cosa state parlando? Per questo la prima seria misura di questo Governo è stata quella di sbloccare concorsi e graduatorie, al fine di dare a Regioni, Province e Comuni una maggiore agilità e rapidità nel reclutamento delle

formazione per militari in servizio, corsi specialistici per formare i nuovi professionisti delle agenzie fiscali e per rafforzarne la capacità funzionale necessaria all'attuazione della riforma tributaria.

a nuove assunzioni in vari Ministeri; abbiamo pensato a supportare le Province interessate dagli eventi alluvionali con nuove assunzioni, oltre autorizzare acquisti di strumenti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile. Abbiamo pensato a introdurre importanti misure per lo sport, come l'esenzione dell'IVA per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI: questa è una misura importante perché impatta sulle famiglie e sui costi per sostenere le attività sportive. Queste sono le misure le risposte di questo Governo e non le vostre chiacchiere. Abbiamo realizzato interventi importanti nel mondo della scuola per dare le risposte che i Governi precedenti hanno lasciato nell'oblio per anni. Abbiamo dato la possibilità di nominare personale ATA necessario a tutte le scuole per poter portare avanti i progetti del PNRR. Abbiamo dato possibilità a tutto il precariato storico del mondo della scuola, attraverso percorsi abilitanti, cose che per anni voi non avete mai fatto. E finalmente adesso i precari delle scuole statali e paritarie possono abilitarsi e ambire ad avere finalmente un contratto a tempo indeterminato.

accade perché questi precari delle scuole paritarie, che per legge sono equiparate dal 2000, non sventolano una tessera di un particolare sindacato?

è che oggi l'Italia è forte di un Governo che, dopo anni di pannicelli caldi, riesce a dare risposte concrete alle problematiche esistenti. Lo fa con provvedimenti seri e non con chiacchiere. Poco Poco fa ho sentito dire che il Governo sul lavoro non ha un'idea. Bene e lo sa perché, signor Presidente? Perché l'idea che aveva il Governo precedente era l'idea di un lavoro-assistenzialismo

che garantisce dignità e futuro ai cittadini italiani e contribuisce al miglioramento della società. Ecco perché abbiamo iniziato con provvedimenti seri, come questo, per eliminare per eliminare situazioni di precarietà con nuove risorse, nuove assunzioni e stabilizzazioni. Sulla pubblica amministrazione, stiamo costruendo le basi per avere un'amministrazione più efficiente, con un rinnovamento serio che parli il linguaggio dell'innovazione, per realizzare quell'ambizioso quell'ambizioso progetto di riforme, che ha l'obiettivo di rendere questa Nazione più moderna, efficiente e orgogliosa di sedere a tutti i tavoli, anche internazionali.

alla sanità e a tutto il pubblico impiego. Per questi motivi, con orgoglio, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia

per portare all'attenzione dell'Assemblea e per richiedere al Governo un'informativa su un fatto di cui oggi parlano alcuni quotidiani, che, se fosse vero,

I giornali di oggi riportano che, a seguito di una denuncia-esposto del ministro Crosetto, sarebbe in corso un'indagine della magistratura riguardante una potenziale centrale di dossieraggio abusivo all'interno della Direzione nazionale antimafia, che avrebbe scavato, negli ultimi anni, nei conti correnti e nelle transazioni finanziarie di centinaia di personaggi noti, tra cui, cito testualmente, politici di primo piano, giornalisti, *manager*, capitani d'industria. Insomma, è una vicenda molto delicata, signor Presidente, e molto particolare. Ci sono degli interrogativi inquietanti che emergono da questa situazione che non riguardano alcuni strati di classe dirigente del nostro Paese, ma libertà fondamentali di tutti i cittadini. *(Applausi)*. Queste ipotesi rievocano Queste ipotesi rievocano pagine non particolarmente edificanti della nostra storia Patria, quando esistevano centrali di dossieraggio che servivano poi a condizionare

sono state innescate da una denuncia esplicita di un membro dell'Esecutivo, quindi siamo in presenza di un fatto istituzionale e politico di assoluta rilevanza su cui chiediamo un'informativa del Governo, un approfondimento dovuto, perché questi temi devono essere messi al centro della nostra attenzione e perché un Parlamento è libero e non può essere condizionato o condizionabile da nessuno. Questa è la base di qualsiasi democrazia.

Borghi, riferirò, come si dice in questi casi.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 votazione nominale con appello. Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no;

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. *(È

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 75. Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15,30 con l'informativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sul reddito di cittadinanza. *(La seduta, sospesa

Signor Presidente, illustri senatori, rendo questa informativa al Senato della Repubblica sul tema del reddito di cittadinanza e delle attività che il Governo sta compiendo per giungere al suo superamento, comprendendo appieno la portata politica dell'argomento. La relazione che vado a illustrare è costituita sulla base di dati analitici, tiene conto delle criticità emerse dall'applicazione del reddito di cittadinanza sin dalla sua introduzione e delinea i passaggi già svolti e quelli in corso di svolgimento per dare piena attuazione alle nuove misure che sono - lo ricordo - legge dello Stato. però dire di più. Il percorso che abbiamo disegnato e che stiamo seguendo con grande attenzione non riguarda solo il semplice superamento di una misura assistenziale e l'introduzione di nuove misure. Direi piuttosto che quest'azione di Governo rappresenta il segno politico di un nuovo approccio culturale che si ispira ai valori del lavoro, così come declinato dalla nostra Costituzione. Vogliamo ribaltare alcune interpretazioni forzate, mosse dalla legittima esigenza di condurre una campagna pregiudizialmente contraria a questa specifica azione del Governo. Vogliamo farlo attraverso i dati e attraverso i fatti

in questo senso è istanza avvertita dal Governo. La nostra sollecitudine e la nostra attenzione sui rischi di marginalità sociale credo siano evidenti e innegabili. Non rinunciamo però a vedere nel lavoro il rimedio vero alla povertà. Pur consapevoli che il bisogno è generalmente multidimensionale, che alla povertà reddituale si accompagnano spesso la povertà educativa e altre forme di deprivazione sociale, continuiamo a credere che il lavoro sia sempre il mezzo migliore per porre rimedio duraturo alle condizioni di indigenza. Accanto a robusti presidi di servizi sociali, occorre definitivamente costruire il sistema di politiche attive del lavoro per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro. Tutti Tutti devono avere il diritto a rendere reversibili i loro percorsi di vita. Nel perimetro delle mie prerogative e responsabilità ministeriali ci sono l'istruzione e la formazione professionale per il contestuale assolvimento dell'obbligo di istruzione e per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali subito spendibili nel mercato del lavoro e delle politiche sociali. Sono consapevole che il mio ruolo è duplice: lavorare per trovare rimedi successivi e per giocare in anticipo. Da una parte, con le politiche sociali dobbiamo costruire soluzioni a problemi vecchi; dall'altra, dobbiamo evitare che se ne aggiungano di nuovi. Le misure disegnate per superare il reddito di cittadinanza possono essere lette alla luce di queste premesse. Abbiamo disegnato due misure proprio perché siamo consapevoli che i bisogni sono multidimensionali, ma anche personali. Dagli stessi dati di monitoraggio si vede che la platea di chi ha beneficiato del reddito di cittadinanza non è omogenea: agli attivabili nel mercato del lavoro si affiancano i fragili, per cui il percorso di inserimento lavorativo arriva solo dopo quello di inclusione sociale. Mi preme ricordare che l'introduzione del reddito di cittadinanza, che ha seguito l'abolizione del reddito d'inclusione (Rei), è avvenuta tra le severe critiche di numerosi componenti di forze politiche che oggi siedono tra i banchi dell'opposizione e che hanno oggi una visione critica delle misure adottate dal Governo. Dopo più di tre anni di operatività, le critiche al reddito di cittadinanza convergono sulla sua inefficacia come misura di politica attiva del lavoro. Il reddito di cittadinanza ha mostrato da subito numerosi aspetti di criticità legati al forte disallineamento tra sostegno monetario e iniziative di attivazione, reso evidente dall'aver iniziato l'erogazione monetaria senza aver prima provveduto a mettere in grado i centri per l'impiego di far fronte ai nuovi compiti loro assegnati sul piano occupazionale. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio sul reddito e la pensione di cittadinanza dell'INPS, nel mese di giugno 2023 i nuclei beneficiari del reddito sono 896.000, mentre i nuclei beneficiari di pensione di cittadinanza sono 115.000, quindi per un totale di un milione di nuclei. Analizzando i nuclei per numero di componenti, emerge che quelli composti da una sola persona a giugno 2023 sono 473.000. Nell'attività di controllo sui percettori di reddito di cittadinanza effettuati dall'Ispettorato nazionale dall'Ispettorato nazionale per il lavoro e dal Nucleo dei carabinieri tutela del lavoro nel periodo dal 2019 al 2023 sono stati intercettati 35.737 fruitori irregolari o con necessità di regolarizzare la posizione. Risultano inoltre, dall'esito dei controlli svolti dalla Guardia di finanza, a decorrere dall'introduzione del reddito di cittadinanza e fino al primo semestre 2023, contributi indebitamente percepiti o indebitamente richiesti per un ammontare di circa 506 milioni di euro. Si rappresenta che il Comando dei carabinieri tutela lavoro ha in corso numerose indagini. A questo ovviamente si aggiunge anche l'attività di controllo che sta effettuando l'INPS. La cancellazione del reddito di cittadinanza dal 1° gennaio 2024 è stata prevista dalla legge di bilancio del 2023 che, nell'ambito di una più ampia riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, ha stabilito che il reddito di cittadinanza avesse una durata massima nel 2023 di sette mesi fino a luglio, per poi essere sostituito da nuove misure, salvo il caso di nucleo con al suo interno persone minorenni o con almeno sessant'anni di età o disabili. La stessa legge di bilancio ha previsto una deroga alla durata di sette mesi per i soggetti non occupabili, ossia non attivabili al lavoro, presi in carico dai servizi sociali prima della scadenza dei sette mesi. Nella scelta del superamento del reddito va inoltre considerato che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, inviando una lettera di costituzione in mora in ragione del fatto che il suo regime di reddito minimo non è in linea con il diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini, soggiornanti di lungo periodo e protezione internazionale. Il cosiddetto decreto lavoro 2023 introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa istituendo l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro. Il nuovo sistema rappresentato dall'assegno di inclusione mira a rendere più fluida la presa in carico da parte dei servizi sociali degli enti territoriali ed è strettamente collegata all'implementazione della misura di supporto per la formazione e per il lavoro legandolo alla reale partecipazione delle persone alla misura di politica attiva del lavoro. Vorrei sottolineare ciò, perché in questo caso il tema è proprio quello dell'effettiva partecipazione. L'SFL rappresenta il naturale rafforzamento della riforma attualmente in corso rappresentata dal programma GOL, azione di riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro. Il principio unificante alla base della riforma delle misure di contrasto alla povertà e uno: chi è attivabile al lavoro deve potersi attivare ed essere preso in carico dai sistemi territoriali per il lavoro finalizzando il percorso alla qualificazione delle competenze e all'inserimento lavorativo. L'assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. L'assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle condizioni che prima citavo (con disabilità, minorenne, con almeno sessant'anni di età, in condizione di svantaggio e inserito in programma di cure e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione). Il supporto per la formazione e il lavoro è la nuova misura di attivazione al lavoro, istituita dal 1° settembre 2023 al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro, di politiche attive del lavoro, comunque denominate. Sono anche compresi tra i progetti il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività. Il percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa presente nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SISL), attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. All'atto della domanda, l'interessato viene informato che, attraverso il SISL, riceverà l'informazione e l'accettazione della sua richiesta per proseguire il percorso di attivazione. A seguito della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il beneficiario è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. Sulla base delle attività proposte, definite nel patto di servizio personalizzato, l'interessato, attraverso il SISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive, comunque denominate, ovvero specifici programmi formativi e progetti utili alla collettività erogati da soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione dai sistemi regionali da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. Nelle misure del supporto per la formazione e il lavoro rientrano anche le azioni del programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori Il beneficiario dell'indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti della partecipazione a queste attività almeno ogni novanta giorni.

l'incentivo occupazionale a favore dei datori di lavoro privati interessati. Gli incentivi previsti si applicano ai percettori del del supporto per la formazione e il lavoro ed è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo SISL, SISL, per consentire appunto un migliore incrocio tra domanda e offerta di lavoro. L'ultimo monitoraggio di GOL evidenzia che la maggior parte delle Regioni ha già attivato i diversi servizi previsti da GOL, servizi per il lavoro e servizi per il lavoro e formazione, con specifici avvisi. Il Ministero, attraverso quattro tavoli tecnici con le Regioni e le Province autonome e la proficua collaborazione a livello politico con gli assessori regionali, ha già condiviso un percorso istituzionale

Si deve precisare che questa è una misura non per il nucleo, ma per il singolo attivabile al lavoro: questo per dire che, laddove abbiamo avuto la contestazione sulla riduzione dell'importo del sostegno economico, non si è tenuto conto di questo aspetto specifico, che si tratta di un sostegno rivolto al singolo e che nei nuclei familiari che hanno più di un soggetto occupabile può essere riconosciuto a tutti quei soggetti che si attivano ed entrano in uno dei percorsi di inclusione lavorativa. Nell'ambito del SISL opera la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, cui il richiedente l'assegno di inclusione o il supporto per la formazione e il lavoro è tenuto a registrarsi per accedere ai benefici. I richiedenti la misura, attraverso la registrazione sulla piattaforma e dopo aver sottoscritto un patto di attivazione digitale, potranno accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, come dicevo prima. Per le finalità descritte, il sistema informativo, attraverso un sistema di interoperabilità, consentirà lo scambio dati tra le diverse piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale del lavoro che vi sono ricomprese: quindi, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, attraverso il quale i servizi per il lavoro comunicano con l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, GePI, la piattaforma per la gestione dei patti per l'inclusione sociale. Il SISL, attualmente nelle fasi conclusive di sviluppo, sarà operativo - lo confermo - dal 1° settembre 2023, così come indicato nel decreto n. Voglio sottolineare che la piattaforma SISL non rappresenta l'ennesimo sistema informativo. Essa ha l'obiettivo di valorizzare le informazioni già presenti nei sistemi in uso dai Comuni e servizi sociali, da una parte, e, dall'altra, l'immenso patrimonio informativo su chi cerca lavoro. Al centro è la condivisione con tutti gli operatori dei servizi per il lavoro e socio assistenziali, che possono concorrere all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo. Con le Regioni e le Province autonome, che ringrazio per la grande e leale collaborazione, siamo tutti impegnati affinché il 1° settembre il sistema sia operativo e si permetta alle persone di richiedere la prima misura prevista in ordine temporale. Per quanto riguarda i dati sui potenziali occupabili, possiamo dire che, in questo momento, la misura del reddito di cittadinanza prevede che la platea dei nuclei familiari beneficiari, sulla base di caratteristiche attinenti l'assenza o no negli ultimi due anni di esperienze lavorative da parte di almeno un componente, individua i nuclei familiari da indirizzare ai servizi sociali e quelli i cui componenti in età attiva vanno invece indirizzati ai centri per l'impiego. Sono esclusi i nuclei beneficiari della pensione di cittadinanza. Per i nuclei tutelati, quelli in condizione di fragilità, ricordo che la misura del reddito di cittadinanza continua fino a dicembre. Per i nuclei cosiddetti occupabili, la durata del reddito di cittadinanza è di sette mesi e, comunque, non oltre il 31 dicembre del 2023. Comunque - come ricordavo prima - il limite temporale dei sette mesi non si applica ai percettori di reddito di cittadinanza presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. I nuclei familiari indirizzati ai servizi sociali potranno iniziare o proseguire un percorso già avviato e, se presi in carico per la definizione del percorso di inclusione sociale, potranno continuare a ricevere il beneficio fino al 31 dicembre 2023. Nei primi giorni di luglio sono stati comunicati all'INPS 88.000 nuclei presi in carico dai servizi sociali per i quali non si applica il limite dei sette mesi. I componenti dei nuclei indirizzati ai centri per l'impiego, in quanto attivabili al lavoro, potranno accedere, invece, dal 1° di settembre al supporto per la formazione e il lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di realizzare una comunicazione efficace sulle nuove misure, ha istituito un tavolo di lavoro in collaborazione con il Dipartimento informazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e con l'INPS. Il lavoro comune ha permesso di definire un progetto condiviso, che si svilupperà da luglio a dicembre del 2023. La campagna nasce per supportare l'introduzione dei nuovi strumenti, che si pongono come un'evoluzione del reddito di cittadinanza, e mette in evidenza le nuove prospettive di attivazione del Paese che le misure intendono promuovere. In particolare, faccio riferimento al supporto alla formazione e al lavoro, che parte da settembre, e successivamente all'assegno di inclusione. Per supportare l'introduzione delle nuove misure, dal 28 luglio il Ministero del lavoro ha attivato una sezione specifica del proprio sito istituzionale con l'entrata in funzione anche di un *help desk.* 48 del 2023, nell'introdurre le due nuove misure sostitutive del reddito di cittadinanza, ossia l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione, ha definito anche il regime transitorio. Con il messaggio n. 2835 del 31 luglio, l'INPS ha indicato elementi che possono fare chiarezza sulla dinamica in atto per i percettori del reddito di cittadinanza. Nel messaggio si richiama la previsione generale relativa al riconoscimento della misura nel limite delle mensilità enunciate, e comunque entro il 31 dicembre. In secondo luogo, si ricorda che il limite di sette mesi non si applica per coloro che sono stati presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro. A questa platea di non attivabili al lavoro che possono fruire del reddito di cittadinanza oltre il limite di sette mesi, si aggiunge quella composta da nuclei familiari con persone disabili e con altri livelli di fragilità. A ben vedere, fin dalla sua prima modifica prevista dall'ultima legge di bilancio, la fruizione del reddito è stata limitata a chi non si trova in una situazione di particolare fragilità. Per chi invece versa in situazioni di disagio, abbiamo detto qual è l'intervento. La presa in carico di beneficiari di reddito di cittadinanza non attivabili al lavoro da parte dei servizi sociali è possibile fino al prossimo 31 ottobre. I dati a disposizione evidenziano che, dei circa 159.000 nuclei beneficiari sospesi dalla misura per avere esaurito i sette mesi, risultano indirizzati ai Comuni circa 44.000 soggetti e ai centri per l'impiego 112.500 soggetti; dei 44000 indirizzati ai Comuni, 4.000 sono già stati presi in carico e e i Comuni stanno procedendo, attraverso i servizi sociali, alla presa in carico di tutti gli altri soggetti. È importante precisare che, dei 159.000 nuclei interessati dalla sospensione della misura, ben 117.317 sono composti da una singola persona, con incidenze percentuali rispetto al livello territoriale (quindi regionale) di circa il 57 per cento, ad esempio in Campania Sono in corso di emanazione i decreti attuativi del decreto-legge n. 48 del 2023 che consentiranno la piena operatività delle nuove misure nel rispetto della tempistica L'attuazione delle nuove misure di inclusione lavoro è stata al centro dell'ultimo incontro, che si è tenuto il 1° agosto, tra il Ministero e ANPAL, ANPAL Servizi e Regioni, per condividere i prossimi *step* della riforma e cominciare con il nuovo supporto per la formazione e il lavoro. In attesa del 1° settembre, data in entrata in vigore del supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero ha chiarito che i 112.000 nuclei con componenti in età di lavoro compresa fra i diciotto e i cinquantanove anni interessati dalla misura dovranno rivolgersi ai centri per l'impiego. A questo proposito, diverse Regioni hanno già evidenziato di aver avviato una proficua collaborazione con le sedi territoriali dell'INPS per velocizzare tutti i processi. Al fine di velocizzare il più possibile la presa in carico di tutti i potenziali beneficiari delle nuove misure, il Ministero del lavoro sta seguendo con attenzione anche il potenziamento della rete territoriale dei centri per l'impiego, che è un obiettivo che abbiamo in linea con i *focus* del PNRR e del Ministero. In riferimento al coordinamento delle attività svolte dai servizi sociali del Comuni, si evidenzia quanto segue. Dall'entrata in vigore delle nuove norme è stata data tempestiva informazione al gruppo tecnico della rete della protezione e dell'inclusione sociale, composta da rappresentanti del Ministero, delle Regioni e dell'ANCI, convocando diverse riunioni sin dall'emanazione del decreto-legge n. 48 del 2023. A supporto delle attività degli operatori sociali sono stati svolti cinque *webinar* formativi sulla base

Nell'ottica di promuovere il rafforzamento di tutti gli ambiti territoriali sociali, sono inoltre in via di approvazione definitiva apposite linee guida che saranno ulteriormente rafforzate dalle specifiche previsioni introdotte in materia dalla legge delega di riforma per gli anziani non autosufficienti. Ulteriori misure di rafforzamento sono allo studio al fine di estendere la portata del cosiddetto LEPS assistenti sociali e consentirne l'evoluzione in un vero e proprio LEPS *équipe* per la presa in carico sociale. Questo processo sarà concretamente accompagnato e potenziato nell'ambito dell'attività di *capacity building* degli ATS previste con il nuovo programma nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, anche con riferimento alle funzioni gestionali gestionali e organizzative connesse all'integrazione dei sistemi informativi. Avviandomi alla conclusione, tengo a precisare ancora una volta che ad oggi, secondo quanto comunicato dal Ministro dell'interno, non si registrano particolari criticità in ordine a paventate tensioni sociali. Desidero segnalare su questo punto che corre l'obbligo per tutti noi di gestire questa transizione, complessa e articolata, date soprattutto le condizioni di partenza, nello spirito di massima collaborazione istituzionale e di comune responsabilità politica.

Signor Presidente, signora Ministra, devo dire con franchezza che, essendo io un uomo del Novecento che crede che il lavoro nobilita l'uomo, anche perché ho iniziato a fare il fabbro

è questo. Avete scaricato le persone come se fossero un pacco postale. Tutto questo è inaccettabile ed è una vergogna per un Paese come il nostro. Questo è il dato: ripristinare un grande rispetto delle persone.

quell'idea razzista che c'era nei confronti di meridionali. Io sono del Nord, sono nato, cresciuto e vivo lì e conosco benissimo tale cultura, che porta ad avere sempre l'idea che i meridionali non hanno voglia di lavorare. Questo è il dato che vi ha portato a ridurre e a togliere il reddito di cittadinanza. Ed è quello che vi porta a muovervi in questo modo, in particolare contro le singole persone. Questo è l'altro dato: i singoli sono figli di nessuno. Lo ha detto anche lei: il 59 per cento sono singoli. ci doveva spiegare, visto che il decreto lavoro prevede che bisogna fare la formazione, a chi avete fatto la formazione, dove sono i centri per l'impiego,

diritto. Si può essere poveri - ma in questo caso voi non fate la battaglia contro la povertà, ma contro i poveri - e quelli che lo sono, sono indesiderati e quindi vanno emarginati. Questo è il messaggio che voi date; sostanzialmente create una condizione - e lo avete già fatto con il decreto lavoro - costruendo varie categorie

non l'abbiamo chiamata qui per sentire un elenco di cose della durata di mezz'ora, anche perché anche la soglia di attenzione del parlamentare più attento a un certo punto viene raggiunta. Lei avrebbe dovuto venire qui a spiegarci che cosa sta succedendo nel Paese, dopo una decisione presa senza che foste pronti a gestirla. Sul superamento del reddito di cittadinanza sono perfettamente d'accordo: io non ho cambiato idea. Lei diceva che ci sono forze politiche che hanno cambiato idea; si riferiva ai colleghi del PD. Ora non mi faccia spezzare una lancia nei confronti dei colleghi del PD, anche i colleghi della Lega hanno cambiato idea. Ricordiamo benissimo il presidente Conte e il vice presidente Salvini con i cartelli quota 100 e reddito di cittadinanza. Ricordiamo bene quel Governo che aveva sconfitto

che non andavano a rendere questo Paese più prospero. Si dava l'idea che non bisognasse creare ricchezza e prosperità per la collettività, ma che c'era qualcuno che arrivava e, nel momento della stasi, dava il messaggio - mi lasci dire anche moralmente dubbio

Diamo ai nostri giovani il messaggio che non c'è bisogno di sbattersi, di arrangiarsi e di organizzarsi per trovare lavoro e per poter anche realizzare il proprio progetto di vita, perché lavorare significa anche questo. Il messaggio è di non preoccuparsi, perché arriva lo Stato e ci pensa lui.

a concorrervi. Purtroppo le cose stanno così, perché - diciamo la verità - questo è stato presentato come uno strumento di politica attiva del lavoro, ma sappiamo benissimo che soltanto i *navigator* hanno trovato un lavoro grazie al reddito di cittadinanza e nessun altro. Sappiamo che il 70 per cento di chi ha preso il reddito di cittadinanza tre anni fa, lo prende ancora e quindi non c'è stato nessuno sbocco verso un maggior lavoro. Ripeto che si è definanziata la misura industria 4.0 *(Applausi)*, che creava ricchezza per il Paese, per poter finanziare quota 100 e il reddito di cittadinanza: chi lo ha fatto ne porta la responsabilità. Signora Ministra, detto tutto questo e detto che questo istituto andava sicuramente superato, lei non poteva ignorare che l'istituto c'era già. Bisogna capire che le scelte sbagliate della politica non possono essere cancellate con un tratto di penna, non si può tornare al *tamquam non esset*, cioè pensare che basti dire che il reddito di cittadinanza non c'è più per far sì che perché nel frattempo questa sciagurata misura, che appunto ha incoraggiato l'assistenzialismo e non la creazione di lavoro, ha creato delle aspettative. Ministra, quando fa mandare un SMS nel quale dice arrivederci e grazie e poi stamattina dice a RTL 102.5 probabilmente l'SMS era scritto in un modo che non ha dato rassicurazioni e ha creato tensioni, mi viene da chiederle se si rende conto che fa la Ministra di questa Repubblica. Chi ha scritto questo SMS? Chi lo ha mandato? Dov'è il rispetto per le persone? *(Applausi).* Le ripeto: questo è un istituto sbagliato, ma visto che avete fatto una campagna elettorale dicendo che eravate pronti, prima di eliminarlo, voi dovevate... automaticamente)* ...essere sicuri che tutto fosse già perfettamente funzionante, perché l'elenco delle cose che ci ha detto oggi non sappiamo quando, se e come funzioneranno. In un Paese nel quale quella misura aveva già attecchito, il fatto di averla risolta senza avere pronto e operativo uno strumento alternativo *(Applausi)* e con la sciatteria che ha caratterizzato la vostra comunicazione rispetto a gente che vive di quei soldi e di quel reddito, penso sia la dimostrazione di quanto il Governo sia inadeguato a gestire il Paese.

della tanta cattiva propaganda che abbiamo ascoltato. Quello che sta accadendo in queste ore è particolarmente grave, onorevoli colleghi, perché abbiamo i *leader* dei due più grandi partiti di opposizione che soffiano sul fuoco del malessere, fomentando lo scontro sociale *(Applausi. Proteste)* e abbiamo manifestazioni di piazza *ad hoc*, con minacce indirizzate al Presidente del Consiglio, a cui ovviamente va la mia solidarietà e quella di tutto il Gruppo Forza Italia

con toni apocalittici pari ai toni di segno opposto che il Partito Democratico usò nel 2018, quando il reddito di cittadinanza venne approvato. Ce lo ricordiamo bene (io ero in quest'Aula): seppur partendo da posizioni culturali opposte, dicevamo che una misura di quel tipo non avrebbe fatto altro che aumentare il lavoro nero; dicevamo che unificare sotto lo stesso strumento il destino di chi era abile al lavoro e di chi invece non lo era sarebbe stato un grave errore, oltre che molto discriminante; dicevamo che il reddito avrebbe disincentivato culturalmente soprattutto i più giovani dal cercare un posto di lavoro; dicevamo ancora che le maglie erano troppo larghe e che si sarebbero verificati truffe e raggiri ai danni dello Stato e dei contribuenti che pagano le tasse. a distanza di quattro anni non soltanto possiamo dire che queste previsioni si sono rivelate del tutto fondate, ma possiamo rivendicare con orgoglio che Forza Italia non ha mai cambiato idea: la pensavamo così allora e la pensiamo così anche oggi. State cercando di raccontare agli italiani che il Governo dalla sera alla mattina ha deciso di affamare centinaia di migliaia di cittadini; state cercando di raccontare che il sussidio verrà tolto agli italiani che sono impossibilitati a lavorare, ai fragili e alle famiglie disagiate con parenti in condizioni gravi, che devono essere assistiti; state cercando di raccontare agli italiani che il Governo ruba ai poveri per dare ai ricchi. Omettete di dire invece che il reddito di cittadinanza è stato considerato sempre una misura temporanea, con scadenza alla fine del proprio per non rappresentare nel medio termine un disincentivo alla produttività e alla crescita economica. Omettete di dire che il superamento del reddito come lo abbiamo conosciuto finora, cioè a pioggia anche a chi non aveva i requisiti, era già noto dallo scorso dicembre (i famosi sette mesi di proroga della misura). *(Applausi)*. Omettete di dire che in questi mesi grazie all'azione del Governo abbiamo raggiunto il *record* di occupati con un aumento significativo degli occupati stabili. invece, parlano i numeri, non le parole, né la propaganda, né i balconi illuminati a festa. I numeri dunque ci sono e ci dicono che la disoccupazione è in costante calo

Guarda caso, l'anno scorso, malgrado la forte domanda, il settore turistico era andato in *tilt* per la mancanza di personale: non si trovavano camerieri, cuochi o baristi. *(Commenti).* tutto è cambiato e tornano gli stagionali, perché gli ex percettori del reddito che lo hanno preso fino a luglio si sono precipitati a cercare lavoro nei settori della ristorazione e in quello alberghiero, dimostrando quindi di essere stati viziati dal sistema. Omettete di dire che gran parte delle risorse risparmiate grazie al reddito di cittadinanza e al suo superamento sono state utilizzate per tagliare il cuneo fiscale e aumentare gli stipendi proprio alle fasce di reddito più basse. In conclusione, signor Presidente, il dibattito di queste ore appare davvero lunare. Forza Italia invita il Governo ad andare avanti sulla strada tracciata, a predisporre i decreti attuativi per l'attivazione degli strumenti sostitutivi del reddito a riformare gli strumenti per incrociare domanda e offerta di lavoro, a continuare con le politiche di crescita e di sviluppo di nuova occupazione. Vorrei concludere leggendo un biglietto che mi è stato consegnato a mano per strada proprio ieri: «Buongiorno, mi chiamo Claudia, ho venticinque anni, sono laureata in lingue e lavoro in una gelateria. Nonostante molte difficoltà, sono una grande lavoratrice e credo ancora nelle favole. Mi permetto di lasciare il mio numero, se mai potesse aiutarmi per un lavoro.» Lavoro: ecco, di questo hanno bisogno i cittadini, di lavorare. Contestualmente, però, non lasceremo mai soli coloro che per vari

che noi incontriamo per la strada. *(Applausi)*. È per persone come Claudia che non smetteremo mai di impegnarci affinché il lavoro non sia considerato una chimera o una favola, ma una realtà. Questa è la ricetta di Forza Italia da sempre. Questa è la ricetta di questo Governo. Questa è la ricetta su cui gli italiani ci hanno dato fiducia e noi non abbiamo intenzione di tradirli, mi spiace per voi.

per il suo tramite, signor Presidente, vorrei dire che a mio avviso iniziare un intervento tacciando la mia forza politica di clientelismo e terminarlo citando una lettera di una cittadina che cerca lavoro dando in mano un biglietto a un parlamentare forse non è proprio il modo più congruo di iniziare e finire il proprio intervento e non va citato come modello. Non avrei mai pensato di iniziare un intervento dicendo che manca la lungimiranza di un *leader* politico che il 21 novembre 2021 disse: i soldi finiti ai furbi sono poca cosa rispetto alla situazione di povertà

è perché lei in dieci mesi non abbia fatto niente. Non c'è la piattaforma: ci sarà forse il primo settembre, ma al momento la piattaforma che doveva risolvere il problema dei centri per l'impiego, del rapporto tra chi cerca lavoro e chi lo offre non c'è. Ha omesso un piccolo dato rispetto ai centri per l'impiego: dal 2019 al 2022, su 6.116 assunzioni possibili per i centri per l'impiego delle Regioni di centrodestra, sono state assunte 1.735 persone, pari al 28 per cento. Alla faccia della grande collaborazione istituzionale delle Regioni che lei ha millantato nel suo intervento. State scaricando sui Comuni il problema dell'assistenza sociale senza fare nulla per potenziarli sul tema dell'assistenza sociale. corsi per riqualificare i lavoratori non c'è traccia: quale sarà il percorso di formazione che dobbiamo far fare alle persone che escono dal mondo del lavoro? Mi sono quindi interrogato sulle ragioni di questo nulla e la risposta è su un quotidiano di oggi:

Io credo che la verità sia molto diversa da questa. Lei, signora Ministro, ha chiuso la sua relazione citando la questione delle tensioni sociali,

Io credo che ci sia un grande problema quando non si riconosce (e non lo fa neanche quella destra italiana che dovrebbe essere una destra sociale) l'esigenza di avere dei diritti sociali universali e non dei favori che il Governo di turno fa a una piccola platea. Questa è la vera questione in ballo. Noi crediamo che sia necessario che lo Stato garantisca i diritti sociali a tutti quelli che ne hanno bisogno, a prescindere dalle scelte politiche di un Governo. Voi avete fatto una narrazione agghiacciante rispetto al tema degli occupabili e dei non occupabili, per poi definire non occupabile un nucleo familiare che ha un figlio

Ma la domanda è questa: se si dice che il reddito di cittadinanza aveva una parte buona, che era quella che riguardava la parte assistenziale, ossia il sostegno al reddito, e una parte delle politiche attive che non funzionava, mi spiega perché siete partiti cancellando la parte che funzionava? È iscritto a parlare il senatore Romeo.

di strumentalizzare o di agitare le tensioni sociali. Quello alla maggioranza è di evitare di mostrare troppo i muscoli su questo tema, pensando che tutti i provvedimenti possono anche essere decisamente perfettibili. Questo perché noi della Lega non siamo né da una parte i custodi dell'integrità del provvedimento - guai a toccarlo perché è come se fosse un *totem* - né siamo, dall'altra, quelli che lo vogliono cancellare,

Proprio come diceva la senatrice Paola Taverna, che fece la dichiarazione di voto quel 27 febbraio del 2019 - lo ricordo perché intervenne dopo di me - il reddito intervenne dopo di me - il reddito di cittadinanza è molto di più di un sostegno economico, molto di più di un sussidio e di puro assistenzialismo, è uno strumento di politica attiva per stare al fianco di persone che chiedono l'opportunità di potersi rimettere in gioco. Ebbene, verificata una legge che con tutte le buone intenzioni vuole raggiungere questo obiettivo,

protestare sotto le sedi dell'INPS in Campania, a Napoli e da altre parti e si è verificato poi che molti di questi avevano altri tipi di lavori in nero e che il reddito di cittadinanza per loro significava arrotondare fondamentalmente lo stipendio. È il classico esempio dei furbi che di fatto

in due parti: l'aiuto ai bisognosi e alla povertà, a persone che per vari motivi non riusciranno mai ad avere accesso al mondo del lavoro (lo garantisce l'articolo 38 della Costituzione: gli inabili al lavoro e quelli che non riescono ad avere mezzi di sussistenza in qualche modo bisogna aiutarli e mantenerli), e l'aiuto all'impiego. Cosa ha fatto il Governo? Mantiene il reddito di cittadinanza per le persone che sono inabili, in difficoltà e non riescono a lavorare (altrimenti diamo messaggi sbagliati alla popolazione) e trasforma quella parte delle politiche attive del lavoro che non ha funzionato in un meccanismo per cui se ti iscrivi al corso di formazione, se dall'altra parte... Per favore, io non vi ho interrotto. Se dall'altra parte ti iscrivi ad un'agenzia per il lavoro, lo Stato garantisce ancora un sostegno, perché sono 350 euro per un certo periodo di tempo.

però ci sono anche tanti quarantenni, quarantacinquenni e cinquantenni che magari hanno rischiato, hanno perso il posto di lavoro o sono in difficoltà per vari motivi. Si potrebbe studiare un'agevolazione che riguardi anche loro, affinché studiando e naturalmente risorse permettendo (questo ormai lo abbiamo capito bene) si riesca a facilitare sempre più il loro inserimento nel mondo del lavoro. Questa è la nostra posizione chiara, di responsabilità ed è questo il modo giusto per affrontare questa tematica.

informativa: non sono 169.000 purtroppo i beneficiari a cui è stato inviato quell'SMS, che - glielo voglio ricordare - recitava in burocratese

169.000, com'era stato comunicato alla stampa dagli organi preposti, ma abbiamo scoperto da lei che sono 159.000 gli SMS. Lei cerca di giustificarlo e dice sì, avete sbagliato. Non dice però «abbiamo sbagliato», ma ci dice in questa relazione che erano 117.000 i nuclei con una sola persona. Dicendo una cosa ancora più grave, sta cercando di dire: scusate, abbiamo sbagliato perché erano nuclei con una sola persona. Erano persone persone che vivono da sole, perché loro la distinzione la fanno anche sulla scelta di vita che hai deciso di fare. *(Applausi)*. Decidono di entrare nella vita delle persone

perché io non conosco nessuno che abbia deciso di nascere povero, abbia deciso di non studiare o abbia deciso di vivere in condizioni drammatiche. Non ne conosco uno. Le garantisco che conosco persone che vogliono uscire da quella condizione e quando non ce la fanno hanno bisogno dello Stato, hanno bisogno che qualcuno tenda loro la mano. Se, signora Ministra, su 25 miliardi - sono i suoi numeri, l'ho seguita nel ragionamento che ha fatto in questa informativa la Guardia di finanza arriva ad aprire dei *dossier* per 500 milioni, stiamo parlando del 2 per cento, allora c'è qualcosa che ha avuto senso *(Applausi)*, perché io non penso che lei, di fronte all'1 o al 2 per cento di pensioni false o di invalidità false, cancelli tutte le pensioni italiane per provare a capire perché ci sono quelli che falsificano alcuni atti. *(Applausi)*. Difende quelli che avevano quel diritto. E voglio dirlo, una volta per tutte, a chi guarda al passato pensando di far propaganda, dimenticando se stesso. Il Partito Democratico nel 2018 non votò per il reddito di cittadinanza. Il Partito Democratico nel 2019, quando si è trattato di renderlo strutturale e di finanziare gli anni successivi al triennio, lo ha votato convintamente nel Governo giallo rosso. E io ho ringraziato Dio che ci fosse il reddito di cittadinanza durante il *lockdown*, perché, se non ci fosse stato, avremmo avuto conflitti sociali veri. *(Applausi)*. Dopodiché, seguo il ragionamento del presidente Romeo: aveva funzionato perfettamente? Aveva funzionato come sussidio. Probabilmente, se avessimo rafforzato il reddito di inclusione, avrebbe funzionato allo stesso modo. Poteva essere migliorato sulle politiche attive del lavoro. Signora Ministra, peccato che lei, sulle politiche attive del lavoro, non abbia tenuto nemmeno un incontro con le organizzazioni sindacali da quando è Ministra. Peccato che sulla precarietà e sul mercato del lavoro non abbia fatto un incontro con le organizzazioni sindacali: uno che fosse uno. Lei ha incontrato le organizzazioni sindacali tre volte: alla faccia della concertazione! Poi, all'improvviso, il Governo di destra, quando parliamo di salario minimo, ci dice che è a favore della contrattazione. Scoprono la centralità delle organizzazioni del lavoro quando si parla di salario minimo, dimenticando che della concertazione loro hanno fatto un *totem* al contrario, come hanno dimostrato con il decreto del 1° maggio. Delle due l'una, signora Ministra: se è centrale quello che pensano i sindacati, io le chiedo di convocare almeno le organizzazioni sindacali, se non vuol convocare le opposizioni, e di aprire un tavolo sulla precarietà sul mercato del lavoro. Chieda per cortesia ai sindaci di che cosa hanno bisogno. Lo chieda agli assistenti sociali, al presidente

Come mangio? Mi aiuti a trovare un posto di lavoro? Vanno lì, senatrice Ronzulli, non dai senatori che passano per strada, perché ci sono gli uffici preposti nei Comuni. se lei farà questo, avrà tutto il nostro sostegno. Viceversa, le chiedo, signora Ministra, così come lo chiediamo a tutto il Governo, di non continuare a non far nulla, con il pretesto di non poter far tutto. Avete, infatti, rinviato tutto a settembre: dall'autonomia al PNRR, dalle riforme sugli enti locali, che tra l'altro avevano anche l'esigenza di discutere di servizi sociali, al reddito di cittadinanza, fino a questa fantomatica piattaforma, che oggi ci ha detto sarà pronta il 1° settembre. Noi ce lo auguriamo. Sappiamo che, ad agosto, queste persone vivranno con il trauma certo di non sapere cosa accadrà tra un mese e con la certezza di non avere un futuro davanti.

senza conoscere i nostri colleghi della sinistra. Ebbene, lei deve tentare, quando fa le informative o le comunicazioni, prima di tutto di parlare come loro vorrebbero che lei parlasse. Ci dicono, infatti, quello che lei dovrebbe dire, quello che lei dovrebbe riferire, come dovrebbe riferirlo, quali numeri dare, che cosa sostanzialmente fare. Il dato abbastanza semplice ed eclatante, però, è che questo provvedimento l'ha voluto un precedente Governo. Questo Governo ha fatto una campagna elettorale con un programma. I partiti della coalizione di questo Governo hanno detto che il reddito di cittadinanza sarebbe stato tolto

compitino, dateci lo spartito di quello che dobbiamo fare *(Applausi)*, di quello che dobbiamo dire, di quello che deve scrivere l'INPS, di quello che deve succedere.

Vediamo anche quello che avete fatto. Avete fatto un provvedimento che in circa quattro anni ha speso 31,5 miliardi: lo

stati utili come forma di sostegno al reddito - poi spiegherò perché sono stati mal spesi anche in questa misura - ma sono stati assolutamente ininfluenti come misura per l'occupazione, come diceva poco fa il collega Romeo, che miracolosamente - beato lui - ricorda quello che ha detto l'allora senatrice Taverna nel 2019. Dicevo, come misura di politica attiva del lavoro questa misura è totalmente fallita e naufragata: non ha trovato lavoro nessuno. L'altra volta vi siete arrabbiati perché vi ho detto che ha trovato lavoro Di Maio ha trovato lavoro Di Maio *(Commenti)*, qualche *navigator* e basta, nessun altro. Quindi come misura di politica attiva non ha funzionato. Se volete, con estrema onestà vi posso dire che anche precedentemente molte delle misure di politica attiva non avevano funzionato. È però un dato dopo dieci mesi del Governo Meloni e del ministro Calderone, l'occupazione cresce, la disoccupazione cala e la domanda di lavoro aumenta. Com'è questa storia? *(Applausi)*.

una metà di questi 31 miliardi li avessimo potuti mettere sulla sanità. Provate a immaginare questo, perché alla fine ogni provvedimento si misura attraverso le alternative possibili, perché è danaro pubblico, non denaro privato che ognuno spende come vuole. Questo provvedimento è stato costoso e inutile; è stato inutile anche dal punto di vista del sostegno al reddito, perché oggi l'INPS ci dice che solo

una parte saranno recuperati perché inabili al lavoro e quindi percepiranno il sostegno previsto; l'altra parte, quella abile al lavoro, cercherà di intercettare le politiche attive del lavoro del Governo e del ministro Calderone per cominciare a lavorare. Di sicuro, non potranno più percepire un reddito per stare a casa.

chi può lavorare da chi non può lavorare. Questo è il messaggio che da oggi in avanti si lancia; chi non può lavorare viene assistito e preso in carico grazie ai provvedimenti messi in campo dal Ministro, chi può lavorare si mette in condizioni di intercettare la domanda con con l'offerta di lavoro. Questo è un messaggio giusto e di buonsenso; un messaggio che caratterizza la visione pragmatica e la concretezza di questo Governo rispetto alle misure ideologiche e dico solo ideologiche, potrei dire elettorali, ma non lo dico - che avete messo in campo voi con il reddito di cittadinanza.

Presidente, la Commissione ha esaurito la valutazione degli emendamenti e consegnato il testo come emendato

nell'auspicio e nella speranza che i pareri richiesti già dalle 15-15,15 siano pervenuti e quindi, ragionevolmente intorno alle 17,30,

Signor Presidente, Governo, colleghi, viste la straordinaria necessità e l'urgenza di fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel costo del mese di luglio, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese, il decreto-legge oggi in esame reca alcune norme transitorie nelle more della definizione di nuove misure emergenziali in materia di trattamenti di integrazione salariale e prevede la promozione di linee guida e procedure concordate tra le parti sociali a tutela dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche. In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 reca in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale una deroga transitoria alla norma che stabilisce l'applicazione di determinati limiti di durata complessiva, anche per ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili. La deroga riguarda i trattamenti relativi alle sospensioni o alle riduzioni dell'attività lavorativa comprese nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023. In virtù di questa deroga transitoria, non è dovuto il contributo addizionale solitamente a carico del datore di lavoro. Le imprese oggetto della deroga sono: le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione di lavorazione di materiali lapidei. Il comma 2 dell'articolo 1 valuta in 8,6 miliardi di euro per il 2023 l'onere derivante e dispone, per la relativa copertura, una corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. L'articolo 2 estende lo stesso trattamento, sempre in via transitoria, ai lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato, nei casi in cui l'attività degli operai agricoli sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto sempre durante il periodo dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023. Il successivo comma 2 ammette i trattamenti in esame in deroga ai limiti di durata relativi al singolo lavoratore e prevede che tali periodi di trattamento siano equiparati ai periodi lavorativi per il computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere previsto dal contratto L'onere derivante dall'articolo 2, valutato in 1,4 milioni di euro per il 2023, trova copertura sempre con una corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. L'articolo 3, nel testo modificato in sede referente, prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute garantiscano la convocazione delle parti sociali, al fine della sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee guida in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a tutela dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche. La riformulazione approvata in sede referente specifica che le linee guida e le procedure suddette riguardano anche la valutazione della correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione. L'articolo 4 differisce al 30 novembre 2023 il versamento del contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico. Il comma 2 proroga dal 31 luglio al 2023 al 30 ottobre 2023 il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di *payback* delle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale. Il comma 2-*bis,* inserito in sede referente, differisce dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine per il versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali dell'importo di un milione di euro, già stanziato al fine dell'erogazione di un contributo in favore di alcune famiglie per i mesi da ottobre a dicembre 2023 a parziale compensazione delle spese per il riscaldamento. In conclusione, vorrei ringraziare il Presidente e tutti i componenti della 10a Commissione, ma soprattutto

l'Assemblea è chiamata a convertire l'ennesimo decreto-legge. Ormai la questione assurge a prassi consolidata: l'iniziativa legislativa ormai appartiene solo al Governo.

Sarà molto soddisfatto un senatore a caso che oggi non c'è (Renzi) il quale, nella sua lunga marcia trionfale verso la maggioranza, potrà apprezzare il frutto di un monocameralismo di fatto che si sta via via sempre consolidando. In questa XIX legislatura si assiste a una rivisitazione o reinterpretazione in chiave peggiorativa della Costituzione, laddove la Camera alla quale viene per prima assegnato il disegno di legge di conversione del decreto-legge provvede ad un compiuto esame, lasciando all'altra il compito di una mera ratifica. Non serve citare i continui moniti del Presidente della Repubblica, ma serve che la maggioranza faccia autocritica sul punto. Per di più, c'è da aggiungere che i tempi di attesa del decreto non risultano compatibili non risultano compatibili con un'attenta analisi del testo da parte del Parlamento. È stato infatti incardinato in Commissione solo l'altro ieri e fissata la scadenza del termine per la presentazione In Commissione questo lo abbiamo fatto presente e c'è stato risposto che vista l'importanza del provvedimento la maggioranza auspicava una rapidità dell'esame anche per dare un segnale di attenzione ai lavoratori e alle imprese. a questo punto occorre segnalare ai colleghi di maggioranza che l'articolo 77 della Costituzione garantisce al Governo, in casi straordinari di necessità e urgenza, l'adozione di provvedimenti

fosse una scusa e la motivazione invece fosse diversa e a questo punto si comprende anche bene con chi ce l'avesse il ministro Crosetto quando ha dichiarato che il Parlamento non lavora: ce l'aveva con i componenti della sua maggioranza. Noi eravamo pronti - voi no a restare e abbiamo presentato un numero consistente di emendamenti pari a 209, proprio per segnalare tale esigenza. Un decreto così importante non può occupare i lavori di Commissione per sole tre ore. In più, segnalo anche in questa sede l'atteggiamento collaborativo che ha avuto il Gruppo, ritirando 194 emendamenti affinché l'esame potesse essere fatto in Aula, presentando solo quelli rimanenti. Purtroppo, però, anche in questo frangente la maggioranza non ha colto la necessità di approvarne almeno qualcuno dei nostri tranne uno. Tuttavia, molti di questi emendamenti, come ci è stato anche detto, risultavano migliorativi del testo, ma non è stato possibile accoglierli. Parliamo di emendamenti volti a conferire carattere permanente alle disposizioni relative, in particolare, agli operai agricoli nei casi di emergenza climatiche, volti a prevedere la sospensione delle attività lavorative in determinati settori in presenza di temperature elevate e ancora la promozione del lavoro agile e abbiamo visto che ormai l'orientamento di questo Governo sul lavoro agile - lo *smart working* - è totalmente negativo. temperature elevate, il divieto di lavoro nei settori agricolo e della pesca, che è stata completamente dimenticata. Per non parlare dell'ingiustificabile esclusione dai benefici dei lavoratori agricoli privi di contratto a tempo indeterminato, che comporta una irragionevole discriminazione a danno della grande maggioranza degli operatori del settore. In più, non sono stati assolutamente menzionati i *rider* e chi è costretto a lavorare in strada come la Polizia urbana e un'altra serie abbastanza vasta di categorie. Non ci sono le coperture: questo è quello che ci è stato detto. Vi sono dei problemi anche sul *timing* dell'entrata in vigore del provvedimento, che infatti è vigente nel momento in cui già da oltre un mese eravamo nel pieno del caldo e se per i lavoratori del settore edile lapideo e delle escavazioni la norma copre un lasso temporale che va dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, per il settore agricolo la medesima disposizione ha effetti inspiegabilmente dal mese successivo. Questo non ce lo spieghiamo. La tutela della salute e della sicurezza rappresenta un elemento fondamentale in qualsiasi ambito lavorativo e deve essere garantita in modo inderogabile. L'esecuzione di mansioni all'aperto, soprattutto durante i periodi di alte temperature, comporta un aumento dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori che i datori di lavoro devono valutare attentamente e che noi abbiamo il dovere di garantire attraverso interventi legislativi specifici. In particolare, è obbligatorio valutare il microclima sia negli ambienti interni che esterni e, se possibile, eliminare o ridurre i rischi attraverso la riorganizzazione degli spazi e degli orari di lavoro. in questo caso l'unica concessione che ci è stata fatta è stata quella di valutare la correlazione tra umidità, temperature e ventilazione. Sul tema sono intervenuti anche gli istituti previdenziali ed assicurativi INPS e Inail, con una comunicazione congiunta del 26 luglio 2022, e nuovamente l'INPS con il messaggio n. 2999 del 28 luglio 2022, per ribadire e chiarire che le imprese che svolgono attività all'aperto (le attività all'aperto sono quelle che abbiamo visto a maggior rischio, in particolare cantieri edili, stradali, lavorazioni sui tetti, facciate e l'utilizzo di materiali che si deteriorano ad alte temperature) possono avanzare domanda di cassa integrazione ordinaria per temperature elevate, con le stesse modalità degli altri eventi meteorologici. Un ulteriore segnale che le organizzazioni di settore hanno evidenziato, ma che è rimasta lettera morta, è quello relativo all'esecuzione e allo svolgimento delle attività all'aperto, come quelle di raccolta e movimentazione della frutta e degli ortaggi, in condizioni di esposizione prolungata al sole in determinate fasce orarie: una disposizione che non avrebbe cambiato una virgola in termini di oneri, ma che avrebbe sprigionato un effetto benefico per la salute e la sicurezza di chi contribuisce a fare il *made in Italy* *(Applausi)* e a dare consistenza alla sovranità alimentare tanto cara al Governo Meloni, concetti validi solo a fasi alternate a quanto pare. A questo punto, un ingenuo potrebbe pensare che il *vulnus* dell'esame in Commissione potrà essere colmato da un compiuto esame in Assemblea, ma sappiamo - e lo vediamo anche oggi dal numero di presenti - che purtroppo non sarà così.

sarà un periodo molto duro per tanti nostri italiani che non potranno andare in vacanza, perché gli avete tolto anche la speranza di un sussidio e oggi l'abbiamo appreso.

Signora Presidente, il provvedimento che stiamo esaminando sarà probabilmente - anzi sicuramente - l'ultimo

L'Italia è tra i Paesi, sicuramente del mondo occidentale e dell'Europa, più vulnerabili per le catastrofi naturali. È per questo che è urgente salvaguardare l'ambiente e salvaguardare anche le conseguenze sociali. Nel mondo le perdite economiche per disastri naturali a livello globale ammontano a 194 miliardi di dollari;

abbiamo visto con l'alluvione in Emilia-Romagna, che in questo momento, per entità, è la terza catastrofe naturale nel mondo: quasi 10 miliardi di dollari. Le ondate di calore estremo e gli incendi hanno provocato la temperatura più alta degli ultimi La manifattura, l'agricoltura, il turismo sono i settori più colpiti. Ecco perché, Presidente, negare la crisi climatica, dilazionando i tempi della transizione ecologica, danneggia il futuro delle imprese e soprattutto la vita delle persone. *(Applausi)*. È per questo che abbiamo così insistito perché non venissero rinviate a non so quando e non so come quelle risorse del PNRR che servivano proprio a questo: alla transizione ecologica, energetica e alla salvaguardia del nostro territorio. Ma per fronteggiare le ondate di calore, così come tutto quello che ne deriva,

Il decreto in oggetto aveva probabilmente questo scopo. Ne è scaturito un provvedimento che - mi permetto di dire - è quantomeno molto parziale. Ciò che è avvenuto in queste settimane a causa dell'emergenza caldo è sotto gli occhi di tutti: Regioni paralizzate, aziende costrette a fermarsi a causa dell'interruzione dell'energia elettrica, incendi. In questo scenario e in queste condizioni, migliaia di lavoratori sono stati costretti a lavorare comunque, esposti a temperature insopportabili, a fenomeni atmosferici incredibili per il periodo, come i nubifragi nelle Regioni del Nord, con la grandine delle dimensioni di un uovo Era necessario che il Governo prendesse l'iniziativa di tutelare questi lavoratori per attuare misure in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ne sono morti di lavoratori per l'ondata di caldo e credo che questo, anche se noi viviamo in questa bell'Aula, con l'aria condizionata, faremmo proprio bene a ricordarcelo. Questo decreto di cui oggi discutiamo è la montagna che ha partorito il topolino. Bene le misure per i lavoratori edili; meno bene quelle per i lavoratori agricoli. Si fa riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici agricoli solo per quelli a tempo indeterminato, sapendo benissimo - tutti noi lo sappiamo - che parliamo di nemmeno il 10 per cento dei lavoratori e delle lavoratrici occupati in agricoltura: il 90

che, quando si lavora in un campo e in una serra a 40-45 gradi percepiti, si muore di infarto anche se si è a tempo determinato e anche se si è un lavoratore stagionale. Sarebbe stata una decisione giusta estendere a tutti questi lavoratori e a tutte queste lavoratrici la possibilità di andare in cassa integrazione, di non compromettere, anche per il futuro, la loro indennità di disoccupazione.

i fattorini e i lavoratori della movimentazione merci e della logistica che, ancora una volta, sono lasciati fuori dall'attenzione del Governo. Con i nostri emendamenti, abbiamo cercato di estendere la platea dei lavoratori e delle lavoratrici interessati dalle conseguenze della emergenza climatica, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Abbiamo trovato porte, orecchie e anche cuore chiusi. Abbiamo chiesto almeno di riattivare, nei settori dove è possibile, lo *smart working*, di evitare il pendolarismo di tanti lavoratori e di tante lavoratrici. Ma neanche questo risultato è stato possibile portare a casa. Non è stato possibile nemmeno per quei lavoratori e quelle lavoratrici che, essendo dipendenti pubblici

Abbiamo bisogno da subito di estendere questi provvedimenti di copertura a tutti i lavoratori interessati. Ma serve anche che il Governo in modo determinato crei le condizioni per un protocollo importante con le forze sociali e datoriali, che metta al centro la sicurezza dei lavoratori e la tutela della salute. Sono stati fatti dei tentativi, ma non si è ancora arrivati a un punto di incontro. Serve ripartire dalla valutazione dei rischi e dalla prevenzione dei fenomeni atmosferici: è l'unica via per evitare di mettere i lavoratori in condizioni di rischio per la propria sicurezza. Chiediamo al Governo di farsi promotore di questa iniziativa, in modo determinato poiché non serve solo un invito; serve credere nelle cose e credere nel confronto con le parti sociali. È necessario che si riparta dai lavoratori, dai diritti, dalle condizioni di lavoro, per ristabilire giuste modalità di lavoro, non sia in condizioni atmosferiche estreme e che non crei condizione di morte, malattia sicuramente grande disagio per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici. *(Applausi)*. Si tratta di una situazione di urgenza

voglio preliminarmente ringraziare il Governo per la sua presenza costante in Commissione, per tutto il contributo che ci ha dato per poter arrivare poi a definire questo provvedimento. Ai ringraziamenti voglio anche associare il Presidente della Commissione e tutti i commissari, perché è evidente che c'è stato un apporto abbastanza generalizzato e comunque collettivo. Tuttavia, alcune precisazioni, cari colleghi, le devo fare. C'è stata una lamentela negli interventi che mi hanno preceduto sul fatto che si è agito d'urgenza. Ma non ci chiediamo: perché agiamo in urgenza? Noi agiamo in urgenza perché prima di questo provvedimento non avete provveduto a fare nulla *(Applausi)*, non abbiamo trovato nulla. quei provvedimenti strutturali che si richiedono adesso, certamente non saremmo stati qui a discutere di un provvedimento di urgenza. Devo dire che noi non ci associamo a quella quella gara di chi va prima al mare, di chi va prima in montagna; non è una gara che ci appassiona e la lasciamo ai bambini, a chi è più bravo. Noi dobbiamo capire se puntualmente siamo presenti nel rispondere ai bisogni della nostra popolazione. Credo che con questo provvedimento si entra nello specifico di alcune categorie di lavoratori che maggiormente soffrono. In politica si può anche dire che sono rimasti fuori quei lavoratori, quegli altri lavoratori e così via; ma in ma in politica si fa una scala di priorità: è stata fatta e su questo concentriamo i nostri interventi.

parlare di emendamenti che introducono la tutela di lavoratori dell'amianto. Penso però, senza disconoscere il valore dell'argomento, che la pertinenza in questo provvedimento

Quando parliamo di questi lavoratori, è giusto che ci sia protezione, ma dobbiamo anche capire che c'è un lavoro che è rivolto a soddisfare bisogni che sono di alimentazione, di assistenza di altre persone,

sono volte, da una parte, a tutelare con la cassa integrazione o con una integrazione salariale i lavoratori che perdono qualcosa per dall'altra parte, non si chiudono le porte a quella che può essere la tutela dei lavoratori. L'elemento più pregnante del provvedimento al l'articolo 3, in cui si parla di un impegno del Ministero del lavoro e delle parti sociali per affrontare con le parti sociali e datoriali, con tutto il mondo che agisce nel settore, linee guida che possano essere utilizzate per affrontare situazioni emergenziali del futuro. È una parte importante che parte importante che doveva essere valorizzata da quella parte politica che sempre ci stona sulla condivisione, sulla compartecipazione e sul confronto con le parti sociali. *(Applausi)*. Ora che lo facciamo noi, nessuno ne parla e si disconosce.

con una risposta di urgenza, è perché non abbiamo trovato prima del nostro insediamento dei provvedimenti strutturali che ci avrebbero sollevati da questo compito. i problemi, i bisogni, le mancanze, tutto quello che non troviamo e, poi, quando diamo una risposta, sia pure di emergenza, ci sentiamo dire che essa non è strutturale. Vivaddio!

Ci avete lasciati orfani di provvedimenti che potevano essere utili già da prima che noi potessimo adottare questo decreto-legge. va quindi un plauso per il lavoro svolto. A tutti noi e al Gruppo Fratelli d'Italia penso vada riconosciuto il merito di essere sempre stati e di essere continuamente accanto, con il Governo Meloni, ai bisogni emergenti, alle urgenze, a chi ha bisogno. Con questo provvedimento ne diamo ampia e concreta dimostrazione. Dichiaro chiusa la discussione generale. Al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere i lavori sul provvedimento, sospendo la seduta fino alle ore 19. *(La seduta, sospesa

impegna il Governo: a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative necessarie

porre alla sua attenzione quello che secondo noi è un grave ritardo: parlo della Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti che attende da un bel po' di tempo la chiusura dei

solo un Gruppo politico, Forza Italia, ancora non ha comunicato i nominativi, bloccando quello che è uno strumento importantissimo per il Parlamento italiano. Pertanto, per fare realmente la lotta ai criminali degli ecoreati e alle ecomafie si continua a ritardare. Sono passati dieci mesi in questa legislatura e posso dire che questa maggioranza è riuscita a battere il *record* delle ultime due legislature. Faccio appello a lei

finestra"). Le posso comunicare - chieda conferma al suo Capogruppo - che nell'ultima Conferenza dei Presidenti di Gruppo ho dato addirittura un *ultimatum* sui tempi con cui bisogna completare. Quindi, siccome l'*ultimatum* è adesso, dico che o adesso, o al primo giorno utile (è la stessa cosa), la prima cosa che farò alla ripresa dei lavori, a settembre, è dire: o ci sono tutti i nomi, o li sceglie il Presidente.

sarò non ristretto, di più: sarò ritirato. Devo dire due cose: intanto faccio mia, non per pigrizia, ma per scelta, la relazione del Presidente della 10a senatore Zaffini. Perlomeno non vi impegno con dichiarazioni scritte. Detto questo, devo affermare sono contro il doppiopesismo, contro gli starnazzamenti che fanno sì che nella sinistra troppi scoprano oggi distonie gravissime del clima e per tanto tempo non hanno fatto un cacchio. *(Applausi)*. Allora, sinceramente mi vergogno un po'.

ha usato il termine «zoppia» come dispregiativo. Io sono stanco di sentire parole come «mongoloidi», «idioti», «spastici»

Potrò sbagliare, potrò dire cose inesatte, ma parolaccia non voglio essere mai e soprattutto non voglio che vengano appellate così personalità, magari sconosciute,

settore agricolo, il provvedimento interviene esclusivamente sui lavoratori a tempo indeterminato, mentre non interviene sugli altri lavoratori e lavoratrici.

Non interviene sui *rider* e su molti lavoratori che in questa situazione di caldo rischiano più di tutti.

ma dall'altra parte. Forse con questo provvedimento con cui siamo dovuti intervenire prendiamo tutti coscienza che i cambiamenti climatici ci sono e non vanno affrontati in termini emergenziali, ma strutturali. Per le ragioni

Ci asteniamo perché certamente ci sono al suo interno delle norme che vanno nella direzione giusta, cioè quella di salvaguardare alcuni settori maggiormente esposti al rischio di emergenza climatica, come i lavoratori dell'edilizia e i lavoratori dell'agricoltura.

e raccogliere l'appello del presidente Mattarella e di altri cinque Capi di Stato, che hanno chiesto che ci sia una tutela e una salvaguardia del sistema climatico. L'Italia è un Paese particolarmente esposto e abbiamo visto quello che è accaduto nei giorni scorsi. Chiedo quindi anche al Governo e al Presidente di adoperarsi in questo senso, anche per avere una legge nazionale sul clima. Infine, chiedo ancora una volta di ripristinare *(Applausi)*, come tutela reale e come momento di prevenzione di una struttura che realmente ha funzionato e che andava davvero a contrastare il dissesto idrogeologico. Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge al nostro esame è stato approvato pochi giorni fa in Consiglio dei ministri, ma è già all'esame del Senato per una rapida approvazione, cui seguirà la definitiva conversione in legge alla Camera. Si tratta di un articolato conciso, ma molto preciso e specifico in materia di trattamenti di integrazione salariale, norme per affrontare un'emergenza temporanea. Quindi è una deroga momentanea alla norma. Viene inoltre estesa, sempre temporalmente, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale ai casi in cui l'attività degli operai agricoli a tempo indeterminato sia ridotta quando sono presenti intemperie stagionali. Noi riteniamo che le disposizioni siano riferite a un periodo emergenziale e che visto che queste emergenze sono ricorrenti, bisognerà intervenire in modo strutturale. Rileviamo ugualmente il fatto che il Governo è intervenuto con un provvedimento immediato - e lo ringraziamo - dando certamente un segnale di attenzione ai lavoratori e alle imprese. Siamo altresì d'accordo sul fatto che queste misure vadano scritte in modo strutturale e studiate dopo l'ascolto attento di tutte le categorie. Ci risulta - e ringraziamo anche di questo - che il Governo sia già impegnato nel confronto con le parti sociali. Al momento riteniamo però importante approvare queste norme, che sono già operative, con il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.

anche più tempo e non con questo clima da gita scolastica che si percepisce questa sera in quest'Aula. Signori, stiamo parlando di un decreto-legge che avete voluto approvare con estrema velocità, vista l'urgenza. Potevamo anche essere d'accordo con voi perché sicuramente la morte di persone sul posto di lavoro a causa delle temperature che si sono raggiunte nel mese di luglio è sicuramente un'urgenza. Non è però un'urgenza imprevedibile, come purtroppo è stato detto in Commissione lavoro, perché di caldo estremo, di cambiamento estremo, di cambiamento climatico e di mutazioni climatiche stiamo parlando da decenni. Forse finalmente avete percepito che sono una realtà. *(Applausi)*. visto che la relatrice Minasi in Aula ha detto che queste temperature erano imprevedibili. Credo che sia stata un'affermazione incauta, visto che tutti quanti le abbiamo previste più volte, tanto che

lavorare in fretta, ma di farlo bene e rendere così davvero un servizio al Paese con delle norme strutturali perché altrimenti l'anno prossimo, a luglio, staremo di nuovo qui a discutere di morti sotto il sole e di interventi da prendere con urgenza. Vi abbiamo chiesto di non dimenticare nessuno perché i *voucher* li avete reintrodotti voi, i lavori stagionali li avete potenziati voi e a questi lavoratori non date nessuna risposta.

non volendo prendere in considerazione neanche qualche emendamento di buonsenso. Ogni tre per due non fate altro che dire che siete a favore della maternità, della famiglia, dell'aumento delle nascite: vi abbiamo chiesto di poter considerare maternità anticipata l'astensione dal lavoro delle lavoratrici sottoposte alle alte temperature e avete detto di no anche a quello: neanche la maternità tutelate con questo provvedimento. Per non parlare, poi, di tutti gli altri lavoratori che avete lasciato fuori - come hanno già detto i miei colleghi - quelli dell'acquacoltura e della pesca totalmente dimenticati. Non c'è poi neanche un passaggio, se volete, su

L'affermazione più frequente del Governo per ogni bocciatura di emendamento è stata quella per cui non ci sarebbero le coperture. Peccato che poi, all'articolo 4 dello stesso provvedimento, spostate e differite in avanti le norme per

i soldi non ci sono, per far restare i soldini nelle tasche di chi già si è arricchito più che a sufficienza, il tempo c'è sempre e c'è l'urgenza in questo provvedimento. Bravi, complimenti. Non mi dilungo oltre, ma penso che siano più che sufficienti le motivazioni. *(Commenti)*. Sì, vi lasciamo andare in vacanza, non vi preoccupate: mentre i lavoratori continuano a morire sotto il sole, voi pensate alle vacanze. Va benissimo, ma intanto il nostro voto

perché ha dimostrato di sapere intervenire tempestivamente sulle varie problematiche che si stanno manifestando in questa legislatura. Lo ha dimostrato il ministro Salvini con il decreto siccità varato ai primi di aprile, quando si poneva il problema delle specifiche misure di attenzione alla resilienza dei sistemi idrici: lotta alle dispersioni idriche, aumento degli invasi e riutilizzo delle acque. Poi purtroppo a maggio si sono verificati gli eventi alluvionali in Emilia-Romagna, Toscana e Marche e il Governo ha dato una risposta subito, in pochi giorni, trovando 2 miliardi. Abbiamo approvato poi il decreto alluvioni, con altri 4,5 miliardi per dare risposte concrete a tutti i settori, compresi i lavoratori autonomi. Poi è arrivato Caronte con le temperature elevatissime, anzi, un Caronte-*bis* rispetto all'anno scorso, ma vorrei sottolineare che nulla con il precedente Governo Draghi e con il ministro Orlando è stato fatto per coloro che lavoravano in strada. Lo stesso è accaduto nel 2016, quando c'era il Niño con il ministro Poletti. il Governo ha dato subito una risposta, a fronte della richiesta dei sindacati: ha aperto un tavolo di confronto e ha emanato questo decreto-legge il 26 luglio, in vigore dal 29 luglio, che ora stiamo convertendo al Senato. Senato. L'aumento delle temperature sull'ambiente di lavoro ha sicuramente un impatto significativo, come l'esaurimento da calore, il colpo di calore e altre malattie legate allo *stress* da calore, comprendendo tutti i lavoratori, compresi quelli del servizio di emergenza

climatica, per quei settori in cui la cassa integrazione non era prevista, come il settore edile, lapideo delle escavazioni, per gli operai agricoli che sono sempre sotto il sole. Quindi è stata prevista la cassa integrazione (CISOA), è stato aperto anche un tavolo di confronto con i sindacati, per la sottoscrizione di linee guida per procedure concordate, ai fini dell'attuazione di un decreto, di un testo unico, per le emergenze del calore. Signor

un lavoratore - era un lavoratore - dei campi di Latina, che il 2 luglio si è sentito male, raccogliendo le melanzane in quegli stessi campi ed è morto dopo due settimane di ricovero in ospedale. Negli stessi giorni, abbiamo saputo che, in un magazzino su cui si stava costruendo il nuovo impianto di Amazon, un lavoratore di settantacinque anni ha lasciato la vita. Non voglio continuare questo elenco, che purtroppo sarebbe molto lungo, né sono partita da qui per dire che c'è una responsabilità di questa maggioranza o di una maggioranza precedente rispetto a queste morti. C'è in verità - vale per tutto il Paese e per tutte le forze politiche - una grande disattenzione al fatto che nel nostro Paese si continua a morire di lavoro e si muore sempre più spesso. Quelle di questo mese sono morti che ci parlano del bisogno di ripensare complessivamente gli strumenti che abbiamo, per proteggere i cittadini e le cittadine, come i lavoratori e le lavoratrici, rispetto ai fatti che la crisi climatica determina. È questa in realtà la pecca prevalente che vediamo nel decreto-legge È quella cioè di non avere utilizzato questa occasione, non dico per costruire la totale revisione del nostro sistema, ma per dire che non è una emergenza, non siamo di fronte ad eventi sporadici, ma siamo di fronte al fatto che abbiamo bisogno di ripensare il nostro modello degli ammortizzatori, il nostro modello delle tutele e come si fa a mettere in protezione, in particolare, tutti i lavoratori e le lavoratrici che lavorano per strada, sotto il sole e nei campi, che sono davvero molti di più di quelli che pensiamo. vorrei dire tramite lei al senatore Zullo, che prima è intervenuto in discussione generale, che non penso che la politica debba scegliere tra quali lavoratori proteggere e quali no. la politica abbia un dovere, che è dare a tutti i lavoratori e le lavoratrici le stesse protezioni e le stesse tutele. *(Applausi)*. È esattamente il fatto che questa stessa protezione e queste stesse tutele mancano

onorevoli colleghi, che avete costruito una risposta sull'unico strumento che è fondamentalmente pagato dalle imprese e dai lavoratori, cioè la cassa integrazione ordinaria. *(Applausi)*. Non avete messo un soldo, neanche uno, per proteggere quei lavoratori che, ad esempio, non essendo lavoratori subordinati - questa è una grande responsabilità di tutti - non hanno alcun accesso alla cassa integrazione ordinaria. Eppure immagino che, anche in quest'Aula, ci sia chi ha ordinato, durante il caldo del mese di luglio, una pizza a casa o una consegna della spesa, non pensando che quel lavoratore stava su una bicicletta, con l'asfalto che si scioglieva e il rischio della propria incolumità E sono i lavoratori delle piattaforme, quelli del futuro, non sono i lavoratori di un tempo che c'era, ma quelli che abbiamo dinanzi a noi. E allora bisognava avere la forza, come si è fatto per esempio durante il Covid e in altre occasioni, di costruire strumenti anche per coloro che non hanno accesso alla cassa integrazione

Siamo disposti a pagare qualunque prezzo per avere il prodotto più fresco possibile in quel momento, anche se tra mezzogiorno e le sei, nelle ore più calde della giornata, bisogna stare nei campi, magari per un *voucher* o un contratto a termine, nell'incertezza di cosa succede il giorno dopo, perché stiamo facendo la raccolta? E allora anche per quei lavoratori e quelle lavoratrici del mondo agricolo non c'è una risposta. E voi lo sapete tutti, perché sappiamo com'è fatto questo Paese, cui i lavoratori a tempo indeterminato in agricoltura sono assolutamente una minoranza; ancor più lo sono durante la stagione estiva, quando in realtà si procede alla raccolta e alla trasformazione attraverso l'uso dei tempi indeterminati. Potrei proseguire e so che non vi farei felici - nell'elencazione dei perché abbiamo bisogno di ricostruire un sistema di tutele che, da un lato, guardi alla crisi climatica e, dall'altro, all'universalità delle tutele per tutti i lavoratori, perché l'idea che si possa continuare a produrre legislazione sul lavoro, che guarda alle singole corporazioni, ai singoli gruppi e ai singoli soggetti, ma non all'insieme del mondo del lavoro, penso che sia una strada assolutamente pericolosa. *(Applausi)*. avendoci detto che potevate spendere pochi soldi rispetto a queste scelte, proprio non capisco perché all'articolo 4 avete deciso e proposto che quel poco che dovevano pagare le aziende energetiche che hanno fatto gli extraprofitti potevamo farglielo pagare un po' dopo; magari forse potevamo farglielo pagare un po' prima e trovare qualche risorsa in più per dare risposte concrete ai lavoratori e alle lavoratrici. Devo dire che, confermando questo nostro giudizio contrario, speriamo però che questo inizio di discussione ci permetta di immaginare che la crisi climatica la riconosciate.

non ci ha particolarmente convinti, perché i rinvii non sono sempre il modo giusto per affrontare il bisogno di dare risposte. *(Applausi)*. Pensiamo che quell'ordine del giorno impegni invece questo Senato e il Governo a fare davvero quella discussione. Fatemi dire

c'è un problema che va affrontato e risolto. Troppo spesso ci sentiamo dire che il Governo vuole confrontarsi, ma poi i provvedimenti arrivano senza quel confronto; ci sentiamo dire che il Governo vuole confrontarsi, ma poi si sceglie la strada della decretazione d'urgenza e dei provvedimenti di breve periodo. Di emergenza in emergenza, nulla sarà più emergenza e ci sarà l'idea di un Paese che non sa che natura ha e che cosa intende affrontare. Forse, dopo qualche mese, bisognerebbe che vi convinceste anche voi che non ci sono solo le emergenze, ma c'è bisogno di un Paese che sappia strutturarsi e rispondere cambiamenti che sono certo epocali, ma che potremmo avere la forza e la capacità di governare positivamente. Se invece continuate a stare nella logica dell'emergenza, credo che dovremmo continuare a renderci conto che non volete dare risposte positive all'insieme dei cittadini e delle cittadine.

come queste che, come ha detto anche la senatrice Camusso poco fa, non vanno nella direzione sbagliata; probabilmente non arrivano fino a dove lei auspicava, ma vanno nella direzione giusta. Comunque non è il primo anno che dobbiamo occuparci delle condizioni dei lavoratori per il caldo. Noi continuiamo a provarci adesso e continueremo - speriamo di farlo insieme - a occuparcene in futuro. Dopodiché devo dire che, per come è stato costruito il decreto-legge, in alcuni interventi ho sentito ancora una volta la necessità, per me sbagliata, di contrapporre il capitale al lavoro. Siamo nel 2023 e credo che l'Italia abbia bisogno di coniugare capitale e lavoro, perché non c'è da stare dalla parte degli degli imprenditori o dei lavori dipendenti; c'è da stare dalla parte dell'Italia, affinché le imprese, grazie ai propri dipendenti, possano produrre più ricchezza in modo che questa possa essere redistribuita *(Applausi),* altrimenti diventa veramente

tetti di spesa. Capite che già il fatto che un'impresa fondamentalmente debba ridare indietro dei soldi alla Regione, un organo su cui giustamente non esercita alcun controllo, è abbastanza bizzarro. Questo è stato un provvedimento semplice per far rientrare molti soldi nelle casse dello Stato, quando il Governo Renzi decise di attuare questa norma pensata dal Governo Monti.

e di dispositivi medici, oltre 500 si trovano in un grande distretto, il polo biomedicale di Mirandola, che ha migliaia di dipendenti. La proroga di oggi non risolve il problema,

il lavoro di parlamentari, incontrando le persone, ma mi auguro che troverete anche occasione per qualche giorno di riposo. Buone vacanze per chi le può fare. *(Applausi).* **Interventi Presidente, abbiamo depositato in quest'Aula una mozione per continuare a chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni per fare in modo che non si spengano le luci, per fare in modo che il Senato e il Parlamento tutto tengano accesi i riflettori e l'attenzione della politica e dell'opinione pubblica sull'omicidio di Giulio Regeni. A più di sette anni di distanza, le circostanze della morte di Giulio, il rapimento e le torture bestiali cui è stato sottoposto per giorni sono una ferita aperta e drammatica per tutti noi, per le coscienze di tutti gli italiani. Non smetteremo di chiedere verità e giustizia. Giulio Regeni è molto più di un volto e di una storia, è un simbolo, rappresenta un'intera generazione di italiani, rappresenta tutti noi e non è possibile dimenticare né fare finta di nulla. Non può essere mai dimenticata la frase pronunciata dalla madre di Giulio dinanzi al suo corpo: «Sul volto di mio figlio ho visto tutto il male del mondo». Giulio non si era mai rassegnato a questo male, perché amava il mondo e l'umanità, da cittadino italiano nel mondo, da giovane studioso. C'è un *murales* molto bello che raffigura Patrick Zaki e Giulio Regeni insieme, abbracciati e sorridenti, con gli occhi piantati nel futuro, nonostante tutto. A maggior ragione dopo la liberazione di Zaki, oggi è il momento per non smettere di chiedere verità e giustizia per Giulio, è il momento di unirci alle parole pronunciate dal presidente Mattarella qualche mese fa: chiediamo che vengano ricostruite le responsabilità. Ci attendiamo una piena risposta da parte delle autorità egiziane. Signor Presidente, i tentativi di depistaggio in questi anni sono stati numerosi e insistiti e sono un ulteriore, volgare oltraggio alla vita di Giulio Regeni. Per questo chiediamo al Governo Meloni di adoperarsi con forza in ogni sede affinché il Governo egiziano collabori finalmente con le autorità giudiziarie italiane per arrivare ad una verità che renda giustizia a Giulio Regeni, alla sua famiglia, all'intero nostro Paese. Il nome di Giulio e quello dell'Italia sono tutt'uno, così come democrazia e rispetto dei diritti inviolabili della persona sono tutt'uno. Raggiungere la verità per Giulio è una questione politica nazionale, riguarda l'idea di Italia che abbiamo e la determinazione a non perdere mai, in nessuna parte, lo Stato di diritto,

che da molti anni ormai rimane privo di risposte concrete.